Le predette Commissioni sono autorizzate a convocarsi a partire da domani per l'esame del suddetto provvedimento. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento, i pareri dovranno essere espressi entro la giornata di giovedì 30 luglio.

oggi si pone un problema che ci fa dire unanimemente che episodi come quello di Viareggio non si devono più verificare.

i due pilastri lungo i quali dobbiamo procedere per riuscire ad andare avanti nell'ambito della sicurezza: la liberalizzazione e il principio del reciproco riconoscimento. Ne deriva quindi che

poter prevedere delle gronde specializzate per il trasporto merci al di fuori degli ambiti urbani. Anche in questo caso si tratta di un auspicio assolutamente condivisibile, ma, per certi versi, di assai difficile realizzazione. Pensiamo, ad esempio, alle aree fortissimamente inurbate a Nord del Po, in cui non di fatto alcuna possibilità di individuare percorsi lontani da abitazioni o da insediamenti industriali. In ogni caso ricordo che,

Governo: a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere, con norma legislativa, di estendere i principi contenuti nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

del contesto regolamentare, organizzativo e gestionale che consenta all'Agenzia italiana per la sicurezza delle ferrovie di meglio assicurare l'esercizio delle missioni e responsabilità legislativamente attribuitele, in linea con le altre agenzie europee». Non si chiede dunque di modificare le altre, ma di recepire questo ordinamento.

è la necessità di prendere atto che il sistema in quanto tale non funziona sul piano della prevenzione, del controllo e della sicurezza e che c'è la necessità di porre in essere tutta una serie di interventi correttivi, sia sul piano normativo che dell'organizzazione, rispetto alla gestione e al funzionamento

della sicurezza del trasporto ferroviario oltre che dare un segnale forte, una risposta importante alle famiglie delle vittime ferroviario di Viareggio e da tutti gli altri disastri. Credo che questa possa essere l'occasione per iniziare un percorso nuovo e diverso in questo settore per affrontare al meglio problemi così seri e gravi per il nostro Paese.

di grande importanza, di grande urgenza. È necessario che tutti insieme ci si impegni seriamente, fortemente e immediatamente per dare risposte concrete e forti alla sicurezza del trasporto ferroviario nel nostro Paese.

*(PD)*. Signora Presidente, è ancora vivo in tutti noi il ricordo del tragico deragliamento del treno merci nella stazione di Viareggio nella notte tra il 29 e il 30 giugno e da allora il bilancio dei morti si è via via aggravato: si contano ormai 28 morti e numerosi sono ancora i feriti ricoverati in gravi condizioni. Al termine del nostro dibattito in Senato, il primo pensiero non può che andare alle vittime e ai loro familiari. Signora Presidente, il dibattito sulle mozioni è stato serio e approfondito, animato dal giusto spirito di una istituzione come la nostra, il Senato, che vuole conoscere fino in fondo i fatti, vuole capire le dinamiche dell'accaduto, vuole individuare le responsabilità dell'evento che ha sconvolto una città, Viareggio, e l'intero Paese. È utile ricordare, come ha già fatto il vice Ministro, le regolamentazioni vigenti sul trasporto delle merci pericolose, che hanno come riferimento il «Libro arancio» dell'ONU. L'obiettivo, che noi condividiamo, è quello di facilitare la libera circolazione delle merci garantendo nel contempo la massima sicurezza. Ma è questo il punto: l'incidente di Viareggio ci interpella proprio sul livello di sicurezza del trasporto merci per ferrovia nel nostro Paese. Se è pur vero che il trasporto su rotaia è mediamente il più sicuro, è altresì evidente che i rischi rimangono considerevolmente alti, poiché almeno il 20 per cento delle merci trasportate rientra nella categoria di merci pericolose. Ogni giorno viaggiano infatti circa 30 convogli con merci pericolose: ammoniaca, benzene, cloro, GPL; queste sono le merci più frequentemente trasportate. Gli incidenti recenti ci obbligano a porre e a porci alcune domande. La prima riguarda l'idoneità della normativa vigente in ordine ai trasporti ferroviari pericolosi: mi sembra che ci sia stata una risposta da parte del Vice ministro rispetto al primo mozione del Gruppo del Partito Democratico sul recepimento della cosiddetta direttiva Seveso anche per il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. Siamo d'accordo anche sulla riformulazione che il Vice ministro ha proposto e riteniamo che questo possa essere un punto fondamentale, un passo in avanti per dare sicurezza al trasporto ferroviario. Il dibattito e le prime verifiche hanno poi sollevato dubbi sul sistema della manutenzione dei vagoni merci; a ciò è preposta l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Ricordo che, in una recente audizione, l'ingegner Chiovelli, direttore dell'Agenzia, ha lamentato lentezze e ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi. Ancora oggi l'Agenzia è drammaticamente sotto organico: sono presenti solo 75 unità di personale, contro una previsione di 300. Credo che il Governo debba fare ogni sforzo perché questo obiettivo di dotare l'Agenzia di un organico idoneo sia raggiunto al più presto. Non si può lesinare, come si è fatto finora, sulle risorse necessarie per far fronte ai compiti che sono stati assegnati dalla legge all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Ricordo inoltre che la Commissione europea ha approvato una modifica della direttiva del 2004 e ha introdotto il cosiddetto ECM, entità incaricata della manutenzione. Ciò determinerà l'obbligo, a partire dal 2010, per ogni vagone, di essere sottoposto a manutenzione da parte di questi enti autorizzati; chiediamo come Partito Democratico di anticipare al 2009 la direttiva sulla responsabilità dell'ECM. Infine, è indispensabile la definizione di una piattaforma informatica europea per lo scambio in tempo reale dei dati relativi all'esercizio e alla manutenzione di tutti i carri ed al trasporto delle merci pericolose. In conclusione, signora Presidente, mi consenta di richiamare la sua attenzione e quella dell'Aula sulla necessità che i dirigenti delle Ferrovie italiane - e aggiungo anche del Governo - si assumano con grande senso di responsabilità il tema della sicurezza ferroviaria in modo ancora più forte di quanto non abbiano fatto fino ad ora. Troppo spesso siamo costretti a chiedere conto di episodi che rivelano falle nei nostri sistemi, troppo spesso ci viene risposto, non senza arroganza, che le nostre ferrovie sono le più sicure nel mondo, negando che esista un problema sicurezza. Il problema esiste e gli incidenti ripetuti di cui stiamo parlando ne sono la prova. Le stesse Ferrovie ne sono consapevoli, se hanno licenziato nel 2007 il responsabile della manutenzione dei carri merci e se nei giorni scorsi è stato sostituito il responsabile della Direzione ingegneria, sicurezza e qualità di sistema. Soprattutto, sul tema della sicurezza ferroviaria sono aperte due inchieste (una a Napoli e una a Civitavecchia) con 10 indagati e 80 società nel mirino. Il sospetto è che 4.000 - sì, quattromila - carri merci destinati alla rottamazione siano ancora in circolazione sulla nostra rete ferroviaria: vere e proprie carrette zombie di proprietà delle Ferrovie dello Stato, riverniciate alla bell'e meglio e riavviate sul mercato con numeri di telaio taroccati. Cosa sa il Governo? Cosa sa il ministro Matteoli? Cosa sa l'ingegner Moretti di tutto ciò? È questa la ragione della rimozione dei dirigenti? Abbiamo diritto di sapere. Hanno diritto di sapere gli italiani. Abbiamo diritto anche di conoscere se siamo di fronte a negligenze, colpevoli negligenze, o ad un sistema organizzato, ad un vero e proprio mercato nero dei carri merci, un mercato a cui sarebbe legata, secondo le indiscrezioni della stampa, una lunga catena di reati, truffe, falsi documentali, false fatturazioni, violazioni delle certificazioni sulla sicurezza. Ce n'é abbastanza per chiedere chiarezza, per chiedere al Governo, al di là delle inchieste della magistratura, di intervenire con decisione e con tempestività, facendo luce sui lati oscuri e preoccupanti emersi in questi ultimi giorni, intervenendo sul *management* delle Ferrovie per chiedere se e quali azioni sono state messe in campo per dissipare tutti i dubbi e tutte le preoccupazioni in ordine alla sicurezza ferroviaria. Lo dobbiamo alle vittime di Viareggio. Lo dobbiamo ai ferrovieri e ai passeggeri, che hanno diritto di lavorare e di viaggiare senza rischiare la vita.

Signora Presidente, anche il Gruppo del PdL, oltre a votare la propria mozione, accogliendo i suggerimenti proposti poco fa dal vice ministro Castelli, favore anche delle altre mozioni, nei confronti delle quali registriamo con viva soddisfazione la convergenza sulle parti dispositive. Con questa raccomandazione e con questo impegno che si richiede al Governo noi riteniamo che la normativa italiana possa fare davvero un salto di qualità che si possano apprestare quelle ulteriori garanzie che sono richieste per evitare che incidenti come quello di Viareggio possano ripetersi. Sul potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, vice ministro Castelli, noi accettiamo la sua correzione, perché ci pare formalmente ineccepibile.

nuova finestra"). Prima di passare alla votazione delle mozioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

G8, signora Presidente.

considerato che siamo favorevoli allo sviluppo della ricerca nel settore delle energie rinnovabili e che riteniamo strategica anche la scelta di investire nel settore del solare a concentrazione. È chiaro che va fatta una precisazione al riguardo, cioè che una politica incentrata solo su questo tipo di intervento rischierebbe di essere deficitaria almeno per due ragioni. La prima è che la forte densità di popolazione nel territorio italiano non permetterebbe una larga diffusione del solare a concentrazione, secondo alcune stime che sono state riportare negli atti al nostro esame. La seconda è che le aziende italiane non sono purtroppo *leader* in questo settore di mercato, per cui questa scelta, se fatta senza un adeguato processo di investimento e di riconversione industriale, rischierebbe di far rimanere fuori dal mercato le piccole e medie imprese italiane. Detto ciò, noi sosteniamo questa iniziativa dei colleghi dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico,

ricorso all'energia nucleare, che è l'unica che può permettere di abbattere costi energetici ed emissioni di CO2 in tempi ragionevoli e quindi non può essere esclusa da alcun mix energetico possibile. Per queste ragioni ribadiamo il voto favorevole su queste mozioni,

Va fatta una distinzione con riferimento alla mozione dei colleghi della Lega, ma purtroppo sul piano dei rapporti fra maggioranza e opposizione avremmo gradito che vi fosse una maggiore attenzione a queste iniziative.

incentivare il settore dell'energia da fonte solare con ciclo termodinamico.

il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.». Questo avveniva il giorno 8 luglio e questa era, a quella data, la posizione della maggioranza e del Governo. Oggi il Governo cambia idea e, in maniera peraltro contraddittoria,

si esprime in questi termini: «...i primi tentativi di realizzare impianti di solare termodinamico anche di consistenti dimensioni... non sono stati persuasivi nei risultati e quindi abbandonati... e pertanto appaiono molto incerte le potenzialità; pertanto, appare economicamente più vantaggioso puntare sulle tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per le quali i costi connessi alla curva di apprendimento risultano prossimi alla combinazione ottimale di efficacia ed efficienza quali, in particolare, le tecnologie del solare fotovoltaico, del consumo di biomasse e dell'eolico» e per concludere: «impegna il Governo: ... a destinare ai suddetti obiettivi», ossia a queste energie alternative, «tutte le possibili risorse, ivi comprese quelle dei fondi non attivati per l'incentivazione di energie non ritenute proficue...» (ossia

è una differenza macroscopica. Come si fa a sostenere entrambe le mozioni? un minimo di attenzione; siamo in un'Aula in cui questi temi hanno una loro importanza, sia pure limitata. Non varremo nulla,

Avevo invitato il senatore D'Alì a rivedere la mozione nella parte in cui impegnava il Governo a tagliare i fondi per il solare termodinamico. Se quella parte viene eliminata, tutte le mozioni (sia quelle che contengono valutazioni critiche che quelle più esaltanti) avranno il medesimo obiettivo, sul quale tutti conveniamo.

tutte le posizioni di questo ramo del Parlamento. Sarebbe un peccato non cogliere questa occasione, mentre il mondo ci sfida proprio su un terreno nel quale abbiamo la *leadership* mondiale in termini di tecnologia.

sono nostre le fabbriche che realizzano all'estero tali impianti; è il nostro genio italiano che ha realizzato le maggiori innovazioni; sono nostre le fabbriche che producono la componentistica. Noi invece non possiamo realizzare, anzi tagliamo i fondi

capofila la Germania, mentre avremmo dovuto esserlo noi, perché il progetto è nostro. Riprendiamo questo treno e questa opportunità. Fate uno sforzo

quale mi onoro di rappresentare il Gruppo. La nostra mozione parla distintamente

centri di ricerca italiani, anche considerando la possibilità della costruzione e sfruttamento di impianti solari termodinamici

far capire che la tecnologia, ad al di là di quel che stiamo facendo, sta andando avanti. Ad esempio, nel mese di giugno di quest'anno alimentato completamente ad energia solare ha varcato le Alpi: è partito da Sion, nel Vallese, ed è atterrato a Torino. Sono passati 99 anni da quando, nel 1910, il primo aeroplano ad energia termica, con un motore a benzina, aveva sorvolato le Alpi, partendo da Briga e atterrando nei pressi nei pressi di Domodossola. Guardate quanta strada ha fatto poi il mondo aeronautico, giungendo al di là non solo delle Alpi, ma degli oceani, con macchine

Continuo anche a dire - e mi rivolgo agli amici della sinistra - che l'ambiente non ha colore, tanto che dichiaro

Abbiamo esitato perché riteniamo che non sia compito nostro, non sia compito del Parlamento, dei Gruppi, né dei singoli parlamentari stabilire quali tecnologie e quali progetti di ricerca e sviluppo siano più meritevoli di essere sviluppati e quali meno. meno. In questo modo, infatti, si invade la sfera dell'autonomia di valutazione dei centri di ricerca, sia pubblici che privati, ed essi, essi solo, devono compiere questa valutazione, mentre alle politiche pubbliche e quindi al Parlamento spetta di fissare gli orientamenti generali e anche la dimensione dello sforzo di sostegno alla ricerca, sia pubblica che privata. Abbiamo esitato, ma poi abbiamo valutato non fosse possibile lasciare che passasse inosservata o rimanesse senza una replica puntuale una mozione come quella proposta dal Popolo della Libertà, nella quale è scritto nero su bianco che l'Italia dovrebbe abbandonare un settore della ricerca, quello del solare termodinamico, che in ogni parte del mondo è considerato tra i più strategici e urgenti, sia in termini ambientali sia sul piano squisitamente economico. Un testo nel quale, devo presumere per motivazioni non proprio nobilissime - soprattutto per dare voce a gelosie un po' miserabili di qualcuno verso uno dei più grandi scienziati italiani, quale è il premio Nobel Carlo Rubbia (che del solare termodinamico è sempre stato un acceso ed aperto sostenitore e che da anni è impegnato perché anche l'Italia sia protagonista nei progetti questa tecnologia) - il PdL sceglie di autoproclamarsi del tutto impropriamente, e se permettete sfidando anche un po' il ridicolo,

che questa innovazione tecnologica, al centro, nel mondo, di rilevantissimi investimenti pubblici e privati, in realtà sarebbe uno spreco di tempo e di denaro. Non è la prima volta che la maggioranza qui in Senato decide di improvvisarsi pseudo-accademia scientifica. È già accaduto con la mozione che nega i cambiamenti climatici, che il Ministro dell'ambiente di un Governo di centrodestra ha dovuto pubblicamente sconfessare; ed è successo con una bozza di risoluzione, poi fortunatamente modificata, in cui si affermava che il nostro Paese dovrebbe chiamarsi fuori dal principale progetto mondiale sulla fusione nucleare. In tutti e tre questi casi, l'esito di queste vostre iniziative - colleghi della maggioranza del PdL - e forse anche l'obiettivo delle vostre iniziative è stato di mettere in discussione le convinzioni, gli orientamenti pressoché unanimi del mondo scientifico, e negli ultimi due casi anche di mettere i bastoni tra le ruote a progetti che vedono protagonista il nostro Paese con i suoi centri di ricerca più autorevoli con i suoi scienziati migliori, con alcune delle sue principali imprese. Rispetto al tema oggetto delle mozioni che stiamo discutendo, per dare supporto a questo che è un atto di vero e proprio sabotaggio della ricerca italiana, voi scrivete che il solare termodinamico non ha futuro. Peccato che secondo le previsioni più caute - non quelle più ottimiste - entro meno di trent'anni saranno installati nel mondo più di 200.000 MW di solare termodinamico (pari a tre volte l'intera potenza elettrica installata in Italia), per una produzione elettrica di quasi 1000 TWh (quattro volte la produzione elettrica italiana). Peccato che solo in Spagna sono già in corso di realizzazione progetti per oltre 10.000 MW di solare termodinamico entro il 2017, quindi entro domani. E peccato che tutti gli analisti del settore concordino che i costi di questa tecnologia sono destinati a scendere rapidamente e sensibilmente, portandosi dagli odierni 8 centesimi di dollaro per kilowattora a meno della metà. Ciò vuol dire che nel mondo, e anche in Italia credo e spero, tra un quarto di secolo il solare termodinamico fornirà più energia, e a costi più bassi considerando gli investimenti iniziali, di quanta ne sia mai venuta e ne verrà mai da una tecnologia molto più vecchia e matura come il nucleare. Al sottosegretario Saglia, che oggi rappresenta qui il Governo e nel cui intervento ho colto un certo imbarazzo nel collegare le argomentazioni in premessa sul tema del solare termodinamico con il parere favorevole dato alla mozione del del PdL, mi rivolgo per chiedergli due banalissimi chiarimenti. Il primo è il seguente: come si conciliano i contenuti della mozione del PdL con gli impegni che il nostro Governo (il vostro Governo), il nostro Ministro dell'ambiente (il vostro Ministro dell'ambiente), hanno assunto anche recentemente nel G8 e prima ancora in sede europea per dare slancio al settore delle rinnovabili, compreso il solare termodinamico. E soprattutto chiedo come tali

a cui il Governo ha dato parere favorevole ed in cui si chiede esattamente il contrario di quello che si chiede nella mozione del Popolo della Libertà, come ha già detto il senatore Li Gotti. Non posso che concordare con lui: un minimo di coerenza rispetto alle vostre premesse, non rispetto a quello che noi chiediamo, sarebbe io credo un buon costume istituzionale. Del resto, anche nelle ultime ore sono venute autorevoli prese di posizione con le quali si manifestano dubbi, perplessità, ed anche un certo sconcerto rispetto ai contenuti della mozione del PdL. Questa mattina il presidente dell'ENEA Paganetto l'ha giudicata singolare. Lei stesso, signor sottosegretario Saglia, partecipando alla presentazione del Rapporto ENEA ha detto che il Governo non intende affatto eliminare gli incentivi al solare termodinamico. Malgrado tutto ciò, il Governo ci ha detto che esprime parere favorevole ad una mozione che, ripeto, afferma il contrario di quello che esso stesso, anche se in maniera secondo me insufficiente, sta cercando di fare, espresso parere favorevole ad una mozione che afferma il contrario di quanto dice la mozione della Lega Nord. che nella mozione della Lega sono scritte le stesse cose che sono scritte in quella del Popolo della Libertà, la contraddizione tra i due documenti, per chiunque sappia leggere l'italiano, è assolutamente evidente. Mi rivolgo allora con un appello ai colleghi della maggioranza ai rappresentanti del Governo, anzitutto perché, invece di battersi (come talvolta, soprattutto qui in Senato fanno) contro l'innovazione energetica provino a fare qualcosa di più perché anche l'Italia si unisca allo sforzo di tutti i Paesi industrializzati verso queste nuove frontiere della ricerca e dello sviluppo che oggi vanno sotto il nome di *green economy* e che nei prossimi decenni avranno la stessa importanza che ebbe negli anni Ottanta e Novanta la rivoluzione informatica.

la smettiate, almeno per una volta, di comportarvi da anti italiani, e facciate quello che in tutto il mondo i Governi, che siano di destra o di sinistra, stanno con difficoltà ed in maniera imperfetta cercando di fare, cioè avvantaggiare i propri Paesi nella corsa verso il futuro, anche verso il futuro dell'economia. Queste sono le ragioni per cui il Gruppo del Partito Democratico, oltre a votare a favore della propria mozione, voterà a favore della mozione presentata dai colleghi dell'Italia dei Valori ed anche di quella presentata dai colleghi della Lega Nord che, ripeto, afferma esattamente il contrario di quella del del PdL. Noi cerchiamo di essere coerenti, e per coerenza non possiamo che votare contro la mozione proposta dal Popolo della Libertà.

e li potrei respingere tutti al mittente; soprattutto in termini di anti italianità avremmo valanghe di argomenti da illustrare nei confronti del PD, come anche sul tema ambientale.

procedere a questo tipo di dichiarazioni.

che riporta una notizia importante che viene da una ricerca scientifica condotta da neozelandesi, quindi al di fuori di questo Parlamento e del sospetto di gelosie (che miseria, senatore Della Seta, parlare di gelosie scientifiche in un dibattito parlamentare).

tutto il dibattito ambientale mondiale ed anche ad influenzare le decisioni dei Governi. Anche il nostro Governo non è esente da questo tipo di suggestioni, nel momento in cui gli si presentano sul tavolo resoconti di possibilità

Abbiamo sollevato un dibattito che sta riscontrando, da alcuni mesi a questa parte, una serie di convergenze sul dubbio relativo

ad annunciare un grande piano di investimento, ma in realtà non parlano della gestione di quegli impianti: parlano della possibilità che le loro industrie forniscano i materiali

sicuramente un interesse industriale dietro la scelta delle energie rinnovabili, che per noi è in senso negativo da questo punto di vista. Non possiamo cedere alle *lobby* industriali di casa nostra o a quelle, molto più forti, del contesto europeo, che vorrebbero che vorrebbero solo fornire impianti, senza accollarsi gli oneri della gestione o il disavanzo tra il costo di produzione ed il valore di mercato dell'energia, continuando ad obbligare i Paesi che devono utilizzare quell'energia ad intervenire

di energia solare. La nostra mozione intende promuovere tutta la ricerca per quanto riguarda le energie rinnovabili. Essa affronta con uno sguardo complessivo l'esigenza di investire in questo settore, ma di farlo

tutte queste considerazioni, contenute nella nostra mozione, non possono che essere condivise da chi ha a cuore un corretto utilizzo delle risorse e del denaro pubblico.

eclatantemente ambiziose e più concretamente utili alla politica energetica del nostro Paese. Non vedo traccia, invece, nelle mozioni del mix energetico che il Parlamento ha approvato proprio nel mese di luglio. Più che seguire alcuni ordini del giorno approvati,

la dipendenza dall'energia tradizionale e, soprattutto, dall'energia proveniente dall'estero si riduca drasticamente al 50 per cento. Pertanto, andare ora ad attivare grandi campi

nuovamente tornare alla dipendenza energetica dall'estero, cioè proprio quello che vogliamo invece evitare con il piano energetico approvato dal Parlamento.

Per cortesia, colleghi, un po' invita a potenziare la presenza strategica nel Paese della tecnologia del solare in tutte le sue applicazioni. Non escludiamo quindi che le applicazioni già finanziate nel settore del termodinamico possano svolgere la loro attività e possano continuare. È chiaro però che se i fondi non sono stati utilizzati pienamente e se le esperienze di altri Paesi non sono esaltanti in questo settore, così come in altri, è giusto che il Governo dia un indirizzo preciso alla sua volontà di sviluppo delle energie rinnovabili.

stessa vuole sostenere nella premessa. Quindi, per una serie di concomitanti ed evidenti contraddizioni fra la premessa e il dispositivo della mozione,

Signora Presidente, vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo qui presenti se non reputino di doversi pronunciare su ciò che sta avvenendo nell'Aula del Senato. Infatti, non avendo nulla da aggiungere alle considerazioni svolte nel merito dai colleghi, e da ultimo dal senatore Della Seta, è assolutamente evidente che le posizioni espresse presentato dalla maggioranza e testé illustrate dal collega D'Alì sono in totale contrasto con le posizioni che il Governo ha manifestato nel vertice del G8 che si è concluso pochi giorni fa.

quella che definisce catastrofiste le posizioni espresse dall'IPCC, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, cui l'Italia

Voi pensate che questo si possa fare, come se il Senato fosse un piccolo ridotto che adotta posizioni scientifiche autonome, o pensate

non è assolutamente corretto quello che lei, senatore Rutelli, ha fatto in questa sede e sono pronto a riaprire il dibattito quando saranno stabiliti tempi congrui su questi argomenti, sui quali abbiamo già dibattuto a lungo e sui quali sicuramente torneremo a dibattere.

stata discrezione della Presidenza aver concesso un minuto al senatore Rutelli. Lei ha dato una risposta che rinvia ad un ulteriore dibattito. Penso che il Governo non debba intervenire.

è molto semplice: il senatore Rutelli ha interrogato il Governo in ordine ad un punto di contraddizione esplicito. Ciascuno di noi ha avuto modo di leggere la mozione presentata dal Popolo della Libertà e ciascuno di noi ha avuto modo di assistere

Ma voi pensate che non crei un principio di contraddizione il fatto che il Senato della Repubblica adotti una mozione con posizioni

situazione assolutamente paradossale, a conferma del fatto che da parte della maggioranza quest'Aula, nel migliore dei casi, viene adoperata come Camera di compensazione di contraddizioni interne alla maggioranza. Sicuramente non le viene attribuito il valore e l'importanza che ha nel nostro sistema costituzionale.

replicare telegraficamente, anche per rispetto nei confronti dei colleghi che hanno partecipato da questa mattina alla discussione, senza

non solo è favorevole agli impegni assunti al G8, ma anzi li sta implementando attraverso una politica volta ad incentivare tutte le fonti energetiche rinnovabili

Ricordo che nella seduta pomeridiana di martedì 21 luglio hanno avuto luogo l'illustrazione e la discussione delle mozioni. Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Mantica, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

favorevole, come pure sul secondo, osservando peraltro che l'indicazione dei 450 milioni di dollari su tre anni forniti dal Governo costituisce una previsione di massima che non comprende gli ammontari, pur rilevanti, dei crediti di aiuto a condizioni agevolate per il settore agricolo e della sicurezza alimentare. Sui capoversi terzo, quarto e

con conseguente riforma del sistema previdenziale e degli ammortizzatori sociali, attraverso la concertazione con le parti sociali, prevedendo l'inserimento di uno stabilizzatore automatico in base al quale l'età pensionabile venga aumentata in relazione all'innalzamento delle prospettive di vita e contemplando al tempo stesso la possibilità di un'estenzione graduale dell'integrazione salariale a tutti i lavoratori;

parere favorevole, a condizione che venga così riformulato: «a rideterminare l'ammontare totale delle risorse destinate agli aiuti pubblici allo sviluppo riallineandole quanto prima in un quadro di compatibilità con la corretta gestione delle finanze pubbliche e del bilancio dello Stato a quanto fissato nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008, nonché alla media europea per poi realizzare l'impegno di raggiungere lo 0,7 per cento del PIL, e a stabilire un programma coerente ed efficiente di cooperazione, evitando la dispersione dell'aiuto, nonché favorendo il coordinamento delle iniziative e dando la priorità all'aiuto verso i Paesi meno avanzati, così da tenere fede agli impegni che l'Italia ha sottoscritto sia a livello europeo che a

a destinare quanto prima, in un quadro di compatibilità con la corretta gestione delle finanze pubbliche e del bilancio dello Stato, i fondi necessari a garantire la partecipazione dell'Italia agli organismi ed ai programmi

il suo articolo di commento al G8. Le valutazioni sul reale esito del confronto fra i Paesi più industrializzati variano di molto, sia fra gli schieramenti politici sia fra i cittadini che leggono la stampa di regime e quelli che invece si informano sui pochi siti e giornali liberi - veramente pochi - che hanno fornito dati seri e comparati. La valutazione varia di molto anche se si guardano i risultati in ottica globale o italiana e se si valutano i benefici che ne hanno tratto gli aquilani in termini di impatto mediatico sull'oggi, oppure in termini di agibilità di case e industrie sul domani e il dopodomani. Dunque, proprio per queste divergenze di valutazione, nell'effettuare la dichiarazione di voto, Presidente e colleghi, voglio fare una riflessione su alcuni punti che esulano dal risultato geopolitico in termini stretti conseguito dai cosiddetti Grandi della terra, per concentrarmi di più sul contesto del G8, cominciando dall'ordine pubblico, dove si scopre che il bilancio è di 11 arrestati, 65 denunciati, tre allontanati dall'Aquila e quattro respinti alla frontiera.

dell'intero bilancio che l'Italia dedica alla lotta alla povertà: 400 milioni di euro a livello di risorse nazionali, più 800 milioni di euro a livello di risorse della Regione Sardegna, contro i miseri 321,8 milioni

che ancora oggi nessuno conosce davvero i conti di questo G8, signora Presidente. Si è parlato di risparmi, ma la confusione delle cifre è totale. è stata spesa in Sardegna. Qualche decina di milioni è stata spesa per le riunioni preparatorie. Altri milioni sono stati spesi all'Aquila per accogliere e proteggere i leader mondiali. Altri soldi ancora sono quelli buttati per le strutture alla Maddalena che non verranno riutilizzate e rimarranno l'ennesimo scheletro architettonico che imbruttisce le nostre coste. Possibile che nel nostro Paese non si possa sapere realmente quanto ci è costato questo G8? Da dove sono stati presi i fondi? A quali altre attività sono stati sottratti?

sarebbero stati più felici di non dover subire i controlli nelle tende, per esempio. Cari colleghi, al di fuori di ogni demagogia o populismo o mediatizzazione del dolore, io credo che, invece che il restauro di qualche monumento, gli aquilani si sarebbero meritati altro: ossia una ricostruzione certa e condivisa. Invece si legge anche oggi sui giornali che la situazione all'Aquila è ancora in alto mare che le abitazioni del nuovo piano case voluto dal Governo non sono sufficienti per tutti i terremotati. Le case diventano a punti, addirittura, e qui cadiamo nel paradossale: solo 4.000 famiglie potranno avere un tetto su 13.000 che dovrebbero essere ospitate. La graduatoria è oltretutto aberrante se si leggono quali sono i requisiti che danno diritto ad avere i punti: cinque punti, il massimo, se li merita chi ha avuto una vittima nel sisma. Sinceramente l'idea della raccolta punti del Governo mi appare insensibile, cinica e cruenta. Inoltre, vi sono paesi ancora del tutto dimenticati, come Castelnuovo di San Pio, che non è stato adottato da nessun leader. Finito il G8, si valuta anche nel complesso l'opportunità di continuare a portare avanti una iniziativa come quella di un *summit* ristretto: in un mondo che cambia rapidamente, la formula G8 è ormai palesemente obsoleta, tant'é che dal G8 si sta rapidamente passando al G20, e ogni anno gli organizzatori di turno sono costretti ad allungare la lista degli invitati. Con questo l'Italia dei Valori, il mio partito, non arriva a dire che il G8 andrebbe abolito, ma se i risultati sono quelli che ha dato forse queste costosissime parate annuali - come le abbiamo definite - dovrebbero essere alleggerite in termini di cerimoniale, così da potere investire su istituzioni internazionali come l'ONU, che possono davvero fare la differenza in termini di obiettivi globali. Ma soprattutto, a 15 giorni dalla conclusione del *summit* internazionale, si tirano le somme. Durante il G8 abbiamo assistito, dai *media* soprattutto televisivi, ad un *reportage* che mostrava le *first ladies* a spasso per Roma a fare *shopping*, mentre tutti mentre tutti ingenuamente aspettavano, davanti ai teleschermi, che "Raiset" ci parlasse dei problemi delle famiglie e della crisi economica: invece, ci si è fermati ai *gossip*, e questo Governo continua a parlare solo di *gossip*. In questo clima più da *gossip* che di sostanza, è dunque naturale che sugli accordi presi ci siano stati, a livello mediatico, confusione e dati parziali. A cominciare dagli aiuti al continente africano, dove è stata buona l'intenzione dei 20 miliardi di aiuti e il partenariato sull'acqua, ma dove rimane anche la circostanza che l'Italia, sia pure nella sua difficile situazione di finanza pubblica, deve sforzarsi di fare materialmente la sua parte, cosa che non fa da due anni. anni. Colleghi, se leggiamo il DPEF e l'assestamento di bilancio, dei soldi necessari per realizzare gli impegni presi non si trova traccia, e neppure nel disegno di rifinanziamento delle missioni internazionali. Se questa maggioranza afferma di voler fermare i flussi di immigrati che arrivano dai Paesi africani e se pensa di farlo respingendo in mare barche di uomini e donne e bambini affamati, disidratati, perseguitati politici, allora essa è formata da una classe politica miope. Sarebbe proprio con adeguati investimenti nei Paesi africani che la soluzione ai flussi diverrebbe stabile e di lungo periodo, oltre che umana e democratica. Se questo importasse ancora a qualcuno!

Ecco allora che tutto si riconduce al problema del pluralismo nell'informazione. Se ci avete attaccato tanto per l'appello che ha fatto il nostro presidente Di Pietro sulla stampa estera durante il G8, un appello che

(dal lodo Alfano alla legge sulle intercettazioni), allora, cari colleghi, avete davvero fatto l'errore di condannare chi denunciava il problema e non il problema stesso. Quello stesso problema che oggi si ripropone con le ultime intercettazioni uscite, che ci parlano di festini, di manie di grandezza del *Premier*, che discetta del G8 non con i suoi parlamentari o con i suoi cittadini, ma con una *escort*! Oggi, con la fusione fra Mediaset e RAI sul digitale, il problema è diventato davvero mostruoso. Ecco perché la nostra mozione presenta una valutazione del G8 diversa da quella di regime, che invece parla solo di risultati straordinari. Se noi mettiamo in luce le ombre è perché la mozione è stata scritta da chi legge e guarda anche altro rispetto all'informazione vendutaci dal nostro *Premier* "mister conflitto di interessi". Tanti cittadini non hanno però né la possibilità, né il tempo, né gli strumenti culturali per fare ciò che gli addetti ai lavori, come noi, hanno potuto fare, ossia una lettura profonda del G8 e dei suoi contenuti al di fuori dei soli *gossip* che le televisioni ci hanno venduto come la sostanza del *summit*. Ecco perché, Presidente, nell'annunciare il voto positivo dell'IdV e nel chiedere anche a voi di votare favorevolmente, vi dico che l'espressione del voto in questo caso non è solo per impegnare il Governo sul G8, ma anche per disimpegnarlo dalla realizzazione di un antidemocratico monopolio dell'informazione a danno di tutti i cittadini.

Il *summit* dell'Aquila è sicuramente stato un successo internazionale tra i più riconosciuti al nostro Governo; un successo che si sintetizza in una serie di impegni profondamente condivisi e di grande valore. ma, poiché alla teoria deve seguire la pratica, agli impegni devono seguire i fatti, alle dichiarazioni devono seguire le azioni. E sia chiaro: non saranno le entità degli stanziamenti a realizzare gli impegni assunti, ma sarà il come tali entità verranno impiegate. Dovranno seguire quindi la strada della vera generosità e della vera umanità. va ricordato ed evidenziato come la cooperazione allo sviluppo non è riconducibile solo ai soldi spesi: provocatoriamente, i *leader* africani ci hanno sfidati, dicendoci: dateci commercio, non dollari! Questa deve essere quindi la strada: accompagnare ogni contributo economico ad opportunità commerciali, e purché sia un commercio basato su principi morali. Il vero nodo, comunque, sarà attuare il cambio da aiuto alimentare a sviluppo rurale, che significa creare le condizioni per poter non solo inviare cibo, ma attraverso il progresso e lo sviluppo creare *in loco* il cibo. Proprio per questo, per la prima volta, è stato creato il Fondo per lo sviluppo rurale, capace di creare le condizioni per far vivere dignitosamente ogni popolo, ma nella propria Patria.

Le conseguenze si toccano con mano: devastazioni ambientali, povertà sempre più dilagante, diritti base calpestati, flussi migratori incontrollati di disperati che si vedono privati del sacrosanto diritto di vivere con dignità nel proprio Paese. Proprio la triste constatazione dell'imponente emergenza data dalle migrazioni di disperati testimonia come in passato qualche cosa non sia funzionato, e che oggi perseverare in tali errori risulterebbe diabolico proprio in contrapposizione al concetto di generosità ed umanità insito negli impegni "abruzzesi". Quindi va riconosciuto e sostenuto il diritto di ogni individuo a poter vivere, progredire e svilupparsi nel proprio Paese partendo anche dagli aiuti internazionali. Quanto da noi oggi promosso, più degnamente lo ha sottolineato Benedetto XVI: il Papa ha sentenziato con alcune frasi ogni concetto e ha saputo indicare la strada per far arrivare a destinazione ogni risultato, anticipando anche temporalmente il lavoro del G8. Per il Santo Padre vi è quindi la promozione dello "sviluppo integrale" dell'uomo, nel senso che non può esservi vero sviluppo senza sviluppo di tutti i popoli e in special modo di quelli più bisognosi. Sicuramente nell'immediato varrà ascoltare quanto auspicato da Papa Benedetto XVI, cioè la ricerca concreta della vera carità quale opposto all'egoismo, del vero sviluppo quale opposto allo sfruttamento, del vero progresso Quindi realmente e concretamente intendiamo impegnare il nostro Governo a proseguire nel cammino intrapreso ricercando con pragmatismo questi tre valori: carità, sviluppo e progresso, affinché attraverso essi si possa consentire ad ogni popolo di vivere con dignità nel proprio Paese senza essere indotto a lasciarlo a prezzo di enormi sofferenze. Il concetto di "aiutare a casa loro", quindi, quale vero segno politica estera. Questi in sintesi gli impegni che con convinzione chiediamo al Governo quest'oggi col consenso dell'Aula. Impegni ambiziosi, destinati evidentemente ad un Paese ambizioso, desideroso di essere considerato quanto equità ed etica potente affinché oggi sia vincente questa giusta potenza sull'ingiusta pre-potenza. **Testo integrale

signor Sottosegretario, penso che la discussione conclusiva sulle mozioni presentate dai diversi Gruppi sull'evento del G8 abbia finito inevitabilmente per essere concentrata prevalentemente non tanto sui contenuti e sui risultati quanto, come accade ormai da molti anni, sulle modalità di svolgimento, sul fatto che non si siano verificati incidenti, che le delegazioni dei Paesi stranieri si siano tutto sommato

(che, come sappiamo, sono vertici informali che si propongono di determinare un punto di vista comune

per gli obiettivi che si propongono alla vigilia. E possiamo dire che nonostante ciascuno di noi faccia uno sforzo - l'hanno fatto anche le mozioni presentate - per cogliere la parte positiva di questo evento che si è svolto in Italia, non possiamo non riconoscere che, leggendo la stampa di oggi, abbiamo l'impressione che forse molte di quelle cose che ci sembravano delle conquiste possono essere rimesse in discussione dal cosiddetto G2, cosiddetto G2, come verrà chiamato d'ora in avanti, cioè dalla sintesi degli interessi fra gli Stati Uniti d'America da una parte e la Cina dall'altra. Chi ha letto la stampa di oggi, per esempio, può cogliere come sul tema del clima sicuramente Obama ha fatto molti passi avanti rispetto a Bush, ma, come ha scritto un importante e autorevole osservatore delle cose internazionali, egli è sempre in conflitto tra ciò che gli dice il cuore e ciò e ciò che invece lo obbligano a fare il pragmatismo e la ragione. Cosa prevarrà nel vertice con la Cina? Il cuore, o la ragione e il pragmatismo, che lo mettono di fronte a un grande Paese, che detiene un quarto del debito che oggi gli Stati Uniti hanno nei confronti del mondo? Mi permetto di avanzare che prevarrà il pragmatismo.

clima. Come sappiamo, l'India e la Cina hanno esplicitamente detto di non essere d'accordo, e se l'India diventa un Paese importante, ancor più lo è la Cina. Quindi, da questo punto di vista, torno al tema di fondo: questi eventi che devono istruire i momenti multilaterali più importanti nei quali si prendono le decisioni, se non risolvono il nodo di come si decide superano il nodo del consenso, per cui un Paese può mettere un veto ed impedire una decisione nell'interesse più generale, rischiano di continuare a svilupparsi richiamando la nostra attenzione sui fatti mondani, sull'efficienza della recettività e così via discorrendo. Penso che dovremo tornare su questo argomento, e su iniziativa del nostro Gruppo proporremo una mozione per affrontare il tema di come l'Italia sta negli organismi multilaterali e di come le sedi che preparano le decisioni degli organismi multilaterali sviluppano l'analisi dei contenuti. Non voglio con questo sminuire alcuni orientamenti - non

Se vogliamo effettivamente risolvere il problema dell'inquinamento, del clima e dell'energia, è da lì che dobbiamo partire, soprattutto quando registriamo differenze così grandi tra i Paesi occidentali sviluppati e i Paesi in ritardo di sviluppo, come quelli dell'Africa.

che già nel vertice di Genova del 2001, su iniziativa del Governo italiano, furono assunte importanti decisioni in quella direzione, ma, come sappiamo, circa dieci anni dopo

accolto il nostro invito ad impegnarsi a fare quelle verifiche e a perseguire quegli obiettivi. Diceva il mio Vice Presidente che di quella mozione dovremmo fare un manifesto e diffonderla nella città della Maddalena.

È balzata alla ribalta del mondo quando l'ammiraglio Nelson, nei primi anni del 1800, vi si rifugiò per circa tre anni con tutta la flotta britannica, facendo la posta alla flotta francese

della base militare americana per missili a testata nucleare. Cito questi due dati per richiamare l'attenzione sul fatto che quando il Governo Prodi

terra, che avevano bisogno di una sorta di risarcimento che poteva certo essere la ribalta mondiale, ma non solo. Ebbene, l'impressione è che al nostro *Premier* questa decisione non sia mai andata bene. Adesso non voglio dire che il terremoto, un evento disastroso e catastrofico, sia stata l'occasione da cogliere per cambiare una decisione. Non lo voglio dire, però consentitemi di esprimere

il messaggio in tempo utile. Penso che questa decisione sia stata presa sicuramente con il buon intento di cogliere un'occasione per dare un aiuto all'Aquila, per la situazione che si è determinata

e dettare possibili terapie. Sotto questo profilo, penso di poter affermare che il vertice dell'Aquila non è stato un insuccesso: diciamolo senza trionfalismi inutili, ma senza altrettanto inutili e talvolta insulse autodenigrazioni. Non vi è stata una

deve essere equilibrato da altrettanto scetticismo, anzi da altrettanto drammatico pessimismo sulle condizioni di decisione della comunità internazionale.

spesso l'uno in funzione dell'altro. Da questo punto di vista, è evidente che il nostro scetticismo su tali vertici deve essere attenuato o quanto meno sfumato.

ha cercato di attenuare le posizioni di Bush (non ho intenzione di riaprire il dibattito sul clima tra il senatore Rutelli ed il senatore D'Alì) perché, senza l'avallo di Pechino, non potranno essere adottate più rigide sanzioni contro Teheran al termine del G20 in programma a settembre a Pittsburgh. Ed allora, presidente Dini, a quelle riunioni delle 8,30 del mattino delle Commissioni esteri congiunte. Noi incontrammo l'ambasciatore Massolo a 24, se non a 48 ore di distanza dal vertice tra Berlusconi ed Obama. Qualcuno di noi - il senatore Perduca ed io stesso avrebbe voluto che il Governo italiano revocasse l'invito non all'Aquila, ma a Trieste rivolto all'Iran. Con eleganza diplomatica l'ambasciatore Massolo ci fece capire che Obama

Nel corso del vertice quello tra Obama e Berlusconi è stato un buon rapporto, perché è stato schietto e sincero; non c'è stato bisogno di demonizzare né Bush, né altri predecessori di Obama per trovare un *feeling* con il Presidente degli Stati Uniti. Senatore Cabras, che cosa ha fatto ieri Obama a Pechino, pensando alle sanzioni di Pittsburgh a settembre? Ha Ha evocato addirittura Nixon nel 1972. Quindi, la retorica giornalistica dei nuovi inizi lascia il tempo che trova in politica internazionale.

Ma soprattutto, senza nessuna volgarità di maniera, riteniamo che questa sia una buona occasione per esprimere un sentimento di gratitudine e di apprezzamento al Governo, alla sobria connessione che c'è stata in questa vicenda fra istituzioni più alte - che non voglio evocare in un'Aula parlamentare - ed il potere esecutivo. Abbiamo dato un buon esempio. Non voglio accentuarne gli aspetti sotto il profilo del trionfalismo, ma penso che lo si possa sobriamente tenere presente nell'apprezzamento che già avevamo espresso proprio in quelle mattine, alle ore 8,30 - per la decisione del Presidente del Consiglio di lasciare La Maddalena e di puntare invece sull'Aquila, non per demagogia, ma perché ci è parso che il mondo fosse attento all'Aquila ed abbia apprezzato quella decisione.

della senatrice Germontani nella discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013**

il DPEF 2010-2013 presenta una revisione alla luce della crisi e delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 il PIL è stimato ridursi del 5,2 per cento rispetto al 4,2 per cento indicato nella relazione unificata.

Un'inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare ad avere un segno positivo con un tasso dello 0,5 Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi molto contenuti.

una lenta ripresa, con una crescita comunque molto più bassa (inferiore al punto percentuale); anche negli anni successivi si evidenzierà un tasso di crescita più basso. Come ha avuto modo di dire l'economista Marco Fortis, nel nostro caso siamo caduti dal primo o dal secondo piano, e comunque ci facciamo male, però altre Nazioni sono cadute dal quarto o dal quinto piano, e dunque si fanno molto più male.

razionali e probabilmente sostenibili nel lungo periodo. Veniamo ora ai dati più importanti relativi all'economia.

dell'acquisto di macchinari e attrezzature proprio a sostegno della domanda di investimenti. Va ricordato poi che gli investimenti hanno un effetto molto positivo sul ciclo generale, anche se con un ritardo di sei-nove mesi. Quindi, è importante partire subito con questa azione di sostegno agli investimenti. In generale, sulla debolezza della domanda hanno influito chiaramente il calo della domanda mondiale, ma anche la stretta creditizia, che purtroppo permane. Nell'audizione

alla caduta delle domande di attività industriali, c'è un dato sintetico del meno 25 per cento di produzione industriale anno su anno, e ciò la dice lunga sull'entità di questa crisi.

È interessante notare come negli oltre dieci anni dal 1995 al 2008 l'Italia ha recuperato in competitività e ha recuperato anche quote di mercato, ma purtroppo oggi subiamo questa crisi in maniera forte. Quindi, è importante l'azione di sostegno al sistema delle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi,

Il dato di sintesi è che per il 2009 sono previsti quasi 76 miliardi di euro di interessi, con un costo medio del 4,6.

è abbastanza scontato e, quindi, anche il servizio del debito potrebbe crescere più di quanto si prevede. Della spesa abbiamo detto: purtroppo questa si mantiene rigida in quasi tutte le sue componenti. Passando ad un'analisi delle entrate, anche per dare una risposta al dibattito emerso già in sede di assestamento e di rendiconto su una presunta

I contributi sociali si mantengono più o meno costanti, con sostanziali piccole variazioni. Questo spiega in larga parte, a nostro avviso, il fatto che si mantenga sugli stessi livelli il dato

della viscosità di alcune imposte (e, in particolare, dei contributi) del calo evidente e scontato del denominatore del PIL, della variazione del *mix* degli acquisti (è evidente che, se siamo in un periodo di crisi, proporzionalmente pesano di più gli acquisti di piccola entità rispetto agli acquisti di grande entità e questo incide sull'IVA). Come

di bilancio, dal punto di vista sia dei conti delle imprese che di finanza pubblica - il DPEF dà anche delle indicazioni sulla priorità di prosecuzione dell'azione di Governo. In quest'ottica il quadro è chiaro: dai dati di finanza pubblica e macroeconomici si evidenzia

ma che purtroppo non vediamo ancora nelle tabelle. Quindi, l'azione riformatrice del Governo dovrebbe portare a questo risultato, altrimenti nel medio periodo i problemi andranno ad acuirsi. Coerentemente il DPEF dà una misura delle azioni riformatrici più importanti da portare avanti in tal senso, anche perché l'altra faccia della medaglia è la tenuta del sistema produttivo. I 720 miliardi di entrate arrivano sostanzialmente dal sistema produttivo privato, quindi è importante che quel settore rimanga in piedi

Intanto quelle che riguardano il settore pubblico, in particolare la pubblica amministrazione e la scuola, dove finalmente si iniziano a premiare il merito e l'efficienza. l'efficienza. Negli ultimi giorni è emerso un dato interessante relativo alla valutazione delle università e ad una diversa distribuzione delle risorse, volta proprio a premiare il merito e l'efficienza. l'efficienza. Questa è, a nostro avviso, la via da perseguire in tutti i settori, anche con maggiore vigore. L'altra riforma a cui il DPEF fa ampio riferimento è quella relativa al codice delle autonomie locali,

a maggior ragione con questi numeri, che la dicono lunga sulla tenuta del sistema - diventa una necessità assoluta. Infatti, se tagliare diventa indispensabile, con il federalismo fiscale quantomeno si riesce a responsabilizzare gli amministratori locali, ad intervenire con criterio sulla spesa, puntando dove più c'è spreco, e a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, che sappiamo essere un problema serio per il nostro Paese, con oltre 100 miliardi di euro all'anno che non entrano nelle casse dello Stato.

che il collega Garavaglia ha poco fa riepilogato, risultano molto più preoccupanti non soltanto delle previsioni elaborate lo scorso anno ed ulteriormente aggiornate, *in peius*, dalla RUEF, ma anche delle più pessimistiche aspettative. I numeri dell'anno in corso e quelli dell'arco temporale previsivo si commentano da sé. Il deficit cresce dal 2,7 al 5,3 per cento per l'anno in corso,

sentire come espressione nelle nostre Aule parlamentari) che non si registrava dal 1991 - quindi, il risultato peggiore da 18 anni a questa parte - e si ricostituisce in senso positivo, ma a livelli molto bassi, a partire dal 2010. Il disavanzo per l'anno corrente peggiora dunque di oltre 38 miliardi di euro, superando gli 81 miliardi in termini assoluti, con un saldo primario ancora più negativo di 43 miliardi. Tali indicazioni sono sostanzialmente coincidenti con quelle elaborate nelle scorse settimane dall'OCSE, dalla Banca d'Italia e dalla Commissione europea, istituzioni che di recente sono state accusate dal Governo italiano di diffondere pessimismo solo perché rendevano noti dati purtroppo molto negativi, che oggi il Governo stesso ufficializza con il DPEF. Tali dati sono ancora più preoccupanti se si considera che la spesa corrente primaria aumenta del 3 per cento del PIL in un anno, un'enormità, raggiungendo il massimo storico del 43,4 per cento, 6 punti in più sul PIL rispetto alla fine degli anni Novanta. La pressione fiscale aumenta dello 0,6

(si tratta del dato più elevato dal 1997, anno nel quale fu introdotta la cosiddetta tassa per l'Europa, poi in parte restituita sulla base dell'impegno assunto con i cittadini). cento, il dato peggiore dal dopoguerra ad oggi, com'è noto, sta tra l'altro producendo effetti devastanti sull'occupazione. Il CNEL stima che il tasso di disoccupazione possa raggiungere a fine anno il 9 con un'ulteriore perdita di posti di lavoro nell'anno in corso fino a 540.000 unità, che diventano 820.000 in termini di ULA Dai dati oggettivi che ho richiamato si ricava la constatazione che tutti gli sforzi di contenimento della spesa e di riconduzione dei saldi di finanza pubblica entro i limiti concordati con la Commissione europea e dentro un quadro di sostenibilità si sono in concreto annullati, e che l'obiettivo del pareggio del bilancio, fissato dal Governo Prodi per il 2011 e confermato lo scorso anno dal Governo Berlusconi, non soltanto è scomparso dall'orizzonte ma è impossibile da cogliere per un periodo lungo e non preventivabile, se la politica di bilancio rimarrà quella delineata nel Documento. Si tratta di un mutamento di scenario di carattere qualitativo, che modifica i "fondamentali" su cui erano stati costruiti gli obiettivi di finanza pubblica da molti anni e ci colloca fuori da qualunque possibilità, nel medio periodo, di rientrare entro i parametri concordati con l'Unione europea prima della crisi. Il volume globale del debito, il livello del *deficit* e della pressione fiscale, la continua ascesa della spesa corrente primaria sono tutti elementi che fanno precipitare il bilancio pubblico italiano ai livelli antecedenti alla metà degli anni '90 e sono destinati a condizionare pesantemente le politiche economiche e di bilancio degli anni futuri. A fronte di tale emergenza, che il Governo ha inteso sin qui minimizzare e ricondurre per intero al ciclo economico recessivo, occorreva una strategia forte di stimolo all'economia e di contestuale correzione dell'andamento tendenziale dei conti a partire dal previsto superamento della fase di recessione.

mentre prevede una riduzione minimale del saldo primario, lo 0,4 per cento del PIL, nel 2011, e di un ulteriore 0,8 per cento sottolineo come il Governo, al pari dell'atteggiamento sostanzialmente rinunciatario e prociclico avuto sulla crisi economica, rinuncia ad un necessario, robusto intervento sui conti pubblici che consenta prima di stabilizzare e poi di ridurre l'andamento della spesa corrente primaria. Non solo: anche i limitati interventi previsti appaiono di difficile realizzazione ed incompleti, cosicché il quadro programmatico proposto, che peraltro viene costruito prendendo a base il quadro tendenziale senza valutare e tener conto delle previsioni a politiche invariate, risulta inattendibile. È sufficiente, al riguardo, richiamare le osservazioni formulate in sede di audizione dalla Corte dei conti. il Governo ha costruito le previsioni per i prossimi anni sulla base di stime della ripresa economica del tutto ottimistiche (crescita dello 0,5 per cento nel prossimo anno e di ben il 2 per cento molto più elevate di quelle adottate dalle altre istituzioni economiche e finanziarie; inoltre, il quadro tendenziale è costruito sul presupposto dell'efficacia dei tagli lineari disposti con il decreto‑legge n. 112 del 2008, che si concentrano, quanto ad entità, proprio nel 2011 (tagli già rivelatisi inefficaci nell'anno corrente), sulla mancata previsione di spese a politiche invariate (quali, ad esempio, quelle necessarie per i rinnovi contrattuali o per taluni investimenti) e di necessità finanziarie già emerse ma non considerate tra gli impegni futuri (quali quelle legate alla spesa sanitaria e agli interventi per il terremoto in Abruzzo). Altro elemento che condiziona fortemente le già modeste previsioni di correzione dei conti è costituito dall'andamento delle entrate, già commentato dal collega Garavaglia. Pur in presenza di una elevatissima pressione fiscale, che si prevede sostanzialmente invariata nel triennio, e dopo aver registrato nell'anno in corso un vero e proprio crollo delle entrate (32 miliardi di euro in meno), si affida la realizzazione degli obiettivi al buon esito della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con una stima di entrata, già prevista in varie disposizioni di legge (da ultimo nel decreto-legge n. 78 del 2009, di cui ci dovremo occupare nei prossimi giorni), di 14 miliardi nel 2010. Il Governo già prevede di recuperare 14 miliardi e su tale dato costruisce il quadro programmatico. Molte ragioni fanno dubitare della realizzabilità di tali obiettivi, considerando anche l'abbandono degli strumenti più efficaci di lotta all'evasione da parte del Governo, il carattere condonistico dello scudo fiscale per i capitali illecitamente esportati all'estero, l'andamento dell'IVA cento nei primi sei mesi del 2009 a fronte di un calo di consumi del 46 per cento), oltre agli effetti dovuti alla ricomposizione dei consumi consumi verso i beni essenziali a più bassa aliquota, gli evidenti sintomi della ripresa dell'evasione. Dunque, alla genericità ed indeterminatezza degli obiettivi di finanza pubblica per i prossimi anni e alla mancata indicazione di precisi strumenti ed interventi correttivi, che rendono peraltro il DPEF non rispettoso delle previsioni dell'articolo 3 della legge di contabilità, si aggiunge un giudizio, che non è solo dell'opposizione ma dei più attenti osservatori e valutatori, di inattendibilità delle previsioni recate nel quadro programmatico. Abbiamo provato in questo anno a dire al Governo e alla maggioranza che la politica economica e di bilancio non era adeguata ad affrontare la più grave recessione dal dopoguerra e che la posizione rinunciataria avrebbe comportato, come è poi avvenuto, effetti sui conti pubblici molto più negativi di quanto si potesse ipotizzare. Il Governo, assumendo il vincolo dell'alto livello del debito e del *deficit*, ha messo in campo diversi ma disorganici interventi anticrisi, muovendosi all'interno dei saldi e quindi sostanzialmente spostando risorse già stanziate da una destinazione all'altra, mobilitando nel complesso risorse molto inferiori a quelle necessarie e a quelle stanziate dai nostri Paesi *partner*:

i tanto declamati interventi anticrisi del Governo. La manovra anticiclica che avevamo proposto lo scorso anno, ovvero mobilitare almeno un punto di PIL, circa 15 miliardi di euro, a favore dei redditi bassi, ammortizzatori per chi non ha protezioni, occupazione e Patto di stabilità interna, prevedendo contestualmente il rientro a partire dal 2010 con misure già individuate sul fronte del contenimento della spesa, alla fine il Governo l'ha fatta ugualmente, ma in una sede inappropriata (l'assestamento), senza organicità e in direzione per lo più casuale, cosicché è facile constatare che gli effetti sui conti sono quelli già registrati per l'anno in corso, mentre gli effetti sull'economia sono tutti da valutare e nessuna seria indicazione di rientro è stata fornita. Pur in un contesto molto peggiorato, continuiamo ad insistere, aggiornandole, sulle nostre proposte. Proponiamo, previo ritiro dell'assestamento e conseguente recupero di un margine finanziario di intervento, un pacchetto di interventi omogeneo ed incisivo, nel brevissimo periodo, in funzione anticiclica, che consenta di intervenire sui redditi bassi, su quelli delle lavoratrici madri e sulla componente variabile delle retribuzioni, di rimuovere i vincoli del Patto di stabilità per i Comuni virtuosi, di concertare con la Cassa depositi e prestiti un intervento per accelerare i pagamenti dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, di ripristinare la piena operatività degli incentivi automatici nel Mezzogiorno e di rendere spendibili le risorse del FAS non ancora utilizzate e già assegnate alle Regioni meridionali, di sostenere con maggior vigore ed efficacia l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese. Proponiamo, inoltre, misure più strutturali, quali la riforma quali la riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, più incisive riforme della pubblica amministrazione, che consentano di razionalizzare la spesa e di recuperare efficienza, un'effettiva riforma dei servizi pubblici locali, misure concrete per lo sviluppo della *green economy* e per il rispetto degli impegni assunti sul clima, l'avvio di una credibile politica per la casa, il riavvio di misure di liberalizzazione, un piano straordinario per il sostegno e il rilancio del Mezzogiorno e il ripristino delle risorse FAS distolte per altre improprie finalità, ed altre più puntuali misure che saranno analiticamente indicate nella nostra proposta di risoluzione. Riteniamo che la riscrittura dell'assestamento, una più incisiva lotta all'evasione e all'elusione fiscale, una diversa misura per il rientro dei capitali senza condoni e con pagamento del dovuto, come hanno fatto gli USA e altri Paesi europei, incisive misure di contenimento selettivo della spesa corrente, anche con la sollecita introduzione dei costi standard e la prosecuzione della politica - che il Governo, a parole, ha ritenuto di dover conservare, ma senza far nulla in questa direzione - della *spending review,* operazioni straordinarie sugli immobili e sul patrimonio pubblici, possano fornire le risorse necessarie per una politica anticrisi più efficace, per attuare le indicate riforme strutturali e per adottare un programma di correzione dell'andamento dei conti pubblici e di rientro dal debito fino al 100 per di cui il nostro Paese ha urgente bisogno. Signor Presidente e signori del Governo, il nostro giudizio sul DPEF e sulla politica economica e di bilancio del Governo è negativo, e le valutazioni per il futuro disegnate nel Documento sono molto preoccupanti. Riteniamo che un'altra politica e un altro DPEF siano possibili ed è ciò che tentiamo di prefigurare con precisione e ponderazione nella nostra proposta di risoluzione. Vogliamo augurarci che, contrariamente a quanto è avvenuto in questo anno, il Governo voglia disporsi all'ascolto e al confronto, anche se è lecito nutrire dubbi su tale volontà. Se ciò non avverrà, noi continueremo a proporre con forza un'altra politica economica, con la convinzione di coltivare gli interessi del Paese e con la facile previsione che i fatti ci daranno ragione.

nel 2009, secondo il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo, essa sarà pari al 43,4 per cento del prodotto interno lordo.

uguale 5,8 punti di prodotto interno lordo in più di spesa corrente primaria. Mal contati, a valori attuali sono 90 miliardi di euro. Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro dell'economia (mi rivolgo a loro per il tramite del vice ministro Vegas), voi che di questi dieci anni ne avete governati sette, voi dovete rispondere a questa banale e precisa domanda: cosa ne avete fatto? Non rispondete, per favore, che li avete usati, almeno in questo ultimo anno, per fare fronte alla crisi: la spesa corrente primaria sale, nell'ultimo anno, di 3 punti secchi di prodotto, ma solo lo 0,7 cioè meno di un quarto di questo aumento, è dovuto alla spesa per ammortizzatori sociali e per il sostegno all'economia. Il resto, la gran parte, due terzi, è semplicemente e banalmente dovuto al fatto che, pur non facendo alcuna manovra espansiva (unico Governo dei Paesi OCSE), non avete tenuto l'evoluzione automatica della spesa sotto controllo. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria di fronte a questa cruda realtà dei fatti circola solo e soltanto rassegnazione. Riassumo così i termini di questa rassegnazione nelle scelte che il Governo fa con questo Documento: primo, non si fanno riforme durante le crisi; secondo, non ci sono spazi per una manovra espansiva nel 2009 corretta da dure e immediate misure di risparmio da far agire quando il ciclo cambierà di segno; terzo, la spesa corrente primaria si potrà ridurre - così ragionate solo - sottolineo: solo - con l'attuazione del federalismo fiscale (cioè a dire: tra sette anni, forse, vedremo qualche risultato); quarto, la pressione fiscale, quella, la programmiamo in aumento di ben 0,6 punti di prodotto nel 2009 («la programmiamo», non «la prevediamo», sono due cose diverse): una pressione fiscale in aumento nel 2009 di più di mezzo punto di prodotto nel corso della più grave recessione che la storia *post* guerra mondiale del nostro Paese conosca, cioè una una politica economica fiscale duramente prociclica come questa non si era mai vista. E non possiamo far altro - aggiunge il DPEF - che tenere quella pressione fiscale al 43 per cento per tutto il periodo di programmazione, fino al 2013 («di programmazione» signor Presidente, non «di previsione»: sono due cose diverse); il quinto, il debito pubblico, infine, risale automaticamente al livello dove stava a metà degli anni '90 e lì resterà, secondo la programmazione del Governo, per tutto il periodo fino al 2013, anche perché - dice il Governo - non abbiamo in animo di adottare misure di valorizzazione del patrimonio pubblico che siano in grado di ridurre più rapidamente il volume globale del debito pubblico. Signori del Governo, voi presentate questo Documento di programmazione economico-finanziaria che adesso ho riassunto e noi saremmo i catastrofisti, quelli che non credono nelle potenzialità del Paese, nella persistenza del suo slancio vitale? La nostra tesi è opposta a quella che voi, col codazzo di commentatori compiacenti e adoranti la "genialità" del Ministro dell'economia, Noi pensiamo che il Paese abbia grandi problemi, ma anche le risorse sufficienti per resistere alla crisi e riproporsi da protagonista nel nuovo ciclo di sviluppo che verrà dopo la crisi: il buon livello del risparmio privato controbilancia l'elevato livello del debito pubblico; il nostro apparato produttivo, specie nella sua componente manufatturiera, è pronto - dopo la dura ristrutturazione del passaggio di secolo ad approfittare di una possibile ripresa dei consumi nell'economia internazionale e della domanda di qualità Italia che può giovarsi dell'esistenza - non so se esserne lieto o no, ma è così - nel mondo di un crescente numero di milionari (in euro, naturalmente); la crisi, infine, indebolisce le posizioni conservatrici di chi si è sempre opposto, sulla base di una logica di tutela neocorporativa dello *status quo*, alle riforme e crea dunque le condizioni la crisi stessa di potenziale consenso politico per fare le riforme. Ma queste potenzialità, che ci sono davvero e che noi vi proponiamo di utilizzare, sono destinate a restare tali, se non viene in campo un progetto consapevole della politica che riduca i fattori di debolezza ed esalti quelli di forza. Questo Documento di programmazione economico-finanziaria - così profondamente intriso di rassegnata impotenza - non è parte di tale progetto. Siamo noi, allora, che vi diciamo: abbiate più fiducia nell'Italia, favorite con le scelte di governo (con i fatti, quindi, non con le polemiche contro gli statistici di tutto il mondo che avete fatto nel corso di queste ultime settimane, in particolare il Ministro dell'economia) la crescita della fiducia degli italiani, quella che gli economisti chiamano il sistema delle aspettative, così importante nell'economia contemporanea. Per farlo, dovreste aprire davvero una diversa fase della vita del vostro Governo: i suoi capisaldi dovrebbero essere specularmente opposti a quelli che hanno contrassegnato questo primo anno di legislatura e che costituiscono l'architrave del Documento di programmazione economico-finanziaria. Primo caposaldo: la crisi è la migliore occasione per fare riforme strutturali. Ne indico tre, a titolo di esempio. una nuova, intensa stagione di liberalizzazioni e di apertura dei mercati chiusi, a partire dal settore energetico - con la separazione proprietaria di SNAM‑Rete gas dall'ENI e dei servizi pubblici locali, per i quali appare preferibile un approccio di settore a quello onnicomprensivo che avete seguito nel decreto n. 112 del 2008 e che ha già fatto fallimento. La seconda: l'adozione di un sistema universale di ammortizzatori sociali che spazzi via gli strumenti gravemente discriminatori tra lavoratori oggi in essere, adottando un moderno sistema di *flex security* di tipo europeo, con tutte le conseguenze del caso, anche sul terreno del diritto del lavoro. La terza: una rivoluzione della giustizia civile che realizzi, a parità di costi e senza modificazioni del diritto sostanziale, ma solo facendo lavorare di più e meglio l'intero sistema, un dimezzamento dei tempi medi del processo italiano, la cui lunghezza spropositata è, tra l'altro, la causa prima della mancanza di investimenti diretti esteri nel nostro Paese. caposaldo, uniti dall'obiettivo di sostenere la produttività e la crescita del sistema economico, da un lato, e, dall'altro, di ridurre al contempo livelli di disuguaglianza, che si sono fatti insostenibili sia sotto il profilo etico che economico. Secondo caposaldo: riprendere subito il controllo dei conti pubblici che voi avete perso, prima di tutto definendo un preciso e verificabile obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria di qui al 2015. Voi nel 2013, con il Documento di programmazione economico-finanziaria, non programmate alcuna manovra correttiva: è un errore grave, che testimonia della totale mancanza di ambizioni che vi sta ispirando. C'è bisogno del contrario: esattamente nel 2013, nel 2014 e nel 2015 la puntuale programmazione di interventi di riduzione della spesa corrente primaria è indispensabile e realistica, se vogliamo recuperare la libertà della nostra politica economica.

se vogliamo che siano efficaci per allora, così da conservare il carattere anticiclico della politica di bilancio. Terzo caposaldo: man mano che si realizzano risultati dal lato della riduzione della spesa corrente, bisogna programmare la riduzione - verso il 40 per cento del prodotto interno lordo nel 2015 - della pressione fiscale; nel frattempo agendo con interventi selettivi per spingere ad un migliore utilizzo dei fattori di crescita, cioè - come dicono gli economisti - per aumentare il cosiddetto prodotto potenziale. *In primis*, per portare a partecipare al mondo del lavoro quei 4 milioni di donne che oggi, a paragone con i grandi *partner* europei, non sono nel mercato del lavoro, ma ne sono fuori, di cui 3 milioni solo nel Mezzogiorno: quei 4 milioni di donne e, in particolare, quei 3 milioni del Mezzogiorno che costituiscono la principale risorsa per lo sviluppo del nostro Sud. E, in secondo luogo, per spostare prelievo - a parità di gettito - dal lavoro, sul quale oggi grava, ai fattori di inquinamento. Quarto caposaldo: un preciso e verificabile obiettivo di riduzione del volume globale del debito, anche attraverso un realistico progetto di valorizzazione del patrimonio pubblico. Anche a questo proposito, il DPEF è rassegnato al peggio (lo definirei così):

Tra il 1995 e il 2004, signor Presidente, abbiamo usato patrimonio pubblico per 11 punti di prodotto interno lordo al fine di ridurre il volume globale del debito; ma il fallimento dal lato del controllo della spesa ci riconsegna un debito pari a quello del 1997. Detto in altre parole: se non ci sarà subito una svolta, la nostra generazione - quella dei *baby boomer* - sarà giudicata come quel nobile che vendeva progressivamente ali del castello per finanziare feste a cui non si divertiva più nessuno. Quinto caposaldo: il ritiro del disegno di legge di assestamento e la sua integrale riscrittura, eliminando ciò che nell'assestamento non ci può stare, cioè l'aumento della spesa e il peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento.

invece di lasciare la qualità della spesa inalterata, come è costretto a fare chi deve ricorrere - come fa il Governo - ad uno strumento improprio come l'assestamento. Nel contesto creato dalle scelte che ho illustrato, una manovra espansiva come questa nel 2009 non allarmerebbe i mercati, non peggiorerebbe il merito di credito, darebbe un piccolo sollievo ad imprese e famiglie e, per questa via, migliorerebbe il sistema delle aspettative. Una politica economica e fiscale di questo tipo crea grandi difficoltà politiche? Certamente sì. Ma è ancora grande il consenso di cui godete ancora nel Paese. Ed è grande la maggioranza su cui potete contare nel Parlamento. Come vi è stato già autorevolmente chiesto: se avete una visione sul futuro del Paese, quando, se non ora, intendete tradurla in impegnative scelte di governo? Quando la legislatura sarà entrata nella sua seconda fase e la vostra luna di miele col Paese sarà soltanto un pallido ricordo? Purtroppo, il vostro Documento di programmazione economico-finanziaria, la vostra rinuncia a tentare di governare la crisi, la vostra rassegnazione ad esserne governati dimostrano che tra i due sentimenti oggi presenti nel Paese - la speranza e la paura - voi avete investito così tanto sul secondo, cioè sulla paura, da restarne prigionieri: facendo leva sulla paura, però, si possono vincere le elezioni, ma si perde la prova del governo

mezzo milione di posti di lavoro a rischio e un tasso di occupazione oscillante tra il 7,9 e l'8,6 per cento. Per dirla più chiaramente, tra 350.000 e 540.000 lavoratori potrebbero perdere il posto di lavoro entro la fine del 2009 e visto il contesto di crescita negativo e le previsioni di un prodotto interno la forchetta della disoccupazione sembrerebbe tendere più verso il 9 per cento che verso il 7 per cento. Gli ultimi dati resi noti dalla Banca d'Italia dicono che la recessione si aggraverà e proseguirà almeno per tutto il 2009 e per il 2010. Oltre 1,2 milioni di lavoratori perderanno il posto di lavoro nel prossimo biennio, con conseguenze sociali devastanti e con un impatto sui consumi che farà da moltiplicatore della crisi. Nel corso del 2009 arriveranno a scadenza più di 2 milioni di contratti di lavoro a termine ed è impossibile prevedere quanti di questi verranno confermati, ma senza dubbio è facile prevedere che la maggioranza di questi non verrà confermata. Nel 2009, pertanto, le liste di disoccupazione rischiano di essere ingrossate soprattutto da lavoratori precari, per i quali non si può neanche parlare di licenziamento, perché semplicemente questi ultimi non vedranno confermato il contratto. Si tratta di lavoratori completamente sprovvisti di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, anche perché al momento non risulta esserci ancora nessun dispositivo attuativo di quegli ammortizzatori in deroga previsti per il 2009. Le risorse che dovevano servire a questo scopo, previste nel decreto-legge n. 185 del 2008, peraltro, sono ancora del tutto bloccate. Il recente rapporto SVIMEZ ha rilevato che nel Meridione, dal 2004 al 2008, i disoccupati impliciti e gli scoraggiati - cioè coloro che hanno rinunciato a cercare un lavoro perché hanno perso davvero ogni speranza sono aumentati di 424.000 unità; e, ancora, che in poco più di 10 anni (fra il 1997 e il 2008) circa 700.000 persone hanno abbandonato il Mezzogiorno e il settore industriale ha subito un calo del PIL del 3,8 per cento. Ma, nonostante ciò, questo DPEF non affronta minimamente il problema della disoccupazione nel Mezzogiorno. Le stime del DPEF 2010-2013 confermano, al di là di ogni accusa di catastrofismo, che la Banca d'Italia, già a fine maggio, aveva visto giusto, indicando, per il 2009, un crollo del PIL di oltre 5 punti percentuali; un ulteriore aumento del debito; l'aumento delle stime sulla disoccupazione, salite in alcune casi a due cifre (il DPEF ci dice infatti che nel solo Mezzogiorno il tasso di disoccupazione del primo trimestre del 2009 è salito al 13,2 che i riflessi della crisi sul mercato del lavoro saranno avvertiti a lungo se il Governo non interverrà con misure incisive: dalla riforma degli ammortizzatori sociali, non più rinviabile, alla riforma del sistema pensionistico. Il DPEF, dopo aver incensato gli interventi adottati dal Governo dall'inizio della XVI legislatura per favorire «il buon funzionamento del mercato del lavoro», sostiene la validità di una serie di norme, in gran parte inserite nel recente decreto-legge n. 78 del 2009, che presentano però numerosi profili di criticità e sono e sono lontane dalle riforme strutturali che sarebbero necessarie per far risollevare l'Italia dall'attuale crisi occupazionale. A pagina 25 del DPEF si legge: «L'utilizzo delle risorse si dispiega in una molteplicità di misure, il cui impatto finanziario si concentra nel triennio 2010-2012, con alcuni effetti di anticipo al 2009. Un pacchetto significativo di interventi mira a sostenere l'occupazione e a rilanciare gli investimenti delle imprese. Le misure specifiche prevedono una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali mediante il rientro anticipato dei lavoratori in cassa integrazione, finalizzato alla formazione, con il riconoscimento di un premio di occupazione alle aziende, in misura equivalente all'indennità spettante al lavoratore cento dello stipendio finanziato dalla CIG, mentre il 20 per cento verrebbe pagato dall'azienda); l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del premio per finalità di auto-impiego; la proroga a 24 mesi del periodo di cassa integrazione per cessazione di attività; l'aumento, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà». Il riferimento specifico è agli articoli del decreto-legge n. 78 del 2009, in cui sono previste le misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento degli ammortizzatori sociali. Devo però rilevare al riguardo, oltre all'irritualità, resa ormai consuetudine, di fare riferimento a norme che in Senato non sono state ancora esaminate né discusse, che tali misure non rappresentano risorse aggiuntive, perché vengono finanziate attraverso la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, presente nell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*,del che tali misure non risolvono il problema della massa di lavoratori dipendenti o parasubordinati che non hanno diritto ad alcun trattamento in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro; che tali misure si risolvono, in buona sostanza, nella proroga della proroga, ovvero nella possibilità concessa ai lavoratori in cassa integrazione di allungare ulteriormente la durata dei trattamenti loro riservati e addirittura riportarli fino al cento per cento del salario precedente frequentando corsi di formazione forniti dalla stessa impresa presso cui operavano. La misura non può certo migliorare le opportunità di impiego di quei lavoratori che sono occupati in quelle tante imprese che non hanno un futuro oltre la crisi e chiuderanno. Rilevo ancora che tali misure, in particolare quelle relative alla cassa integrazione, non sono di immediata applicazione. Infatti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, sarà necessario attendere l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplini le modalità attuative della norma. Nel DPEF, inoltre, non si trova alcun riferimento a politiche strutturali volte a favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia, indispensabili se si vuole innalzare l'età pensionistica delle donne. L'unico riferimento a tale questione è contenuto a pagina 48 del DPEF, dove si legge che «è in fase di avvio un piano di azione sull'occupazione femminile incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro e sulla sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona». Sino ad oggi, però, gli interventi che il Governo Berlusconi ha adottato al riguardo hanno solo peggiorato la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come i tagli all'organico del corpo docente e la detassazione degli straordinari. Una misura, quest'ultima, che certo non può essere applicata alle donne con figli piccoli. Queste scelte hanno provocato l'effetto di bloccare il tasso di partecipazione femminile al 10 per cento. Dobbiamo purtroppo registrare, inoltre, che nel testo si riscontra tutta una serie di falsità ed inesattezze, che non possono essere giustificate all'interno di un Documento di programmazione economico-finanziaria.

che ci sono provvedimenti, tra quelli citati, che in Commissione arrancano e altri che non hanno neanche iniziato il loro *iter*. Avete esautorato il Parlamento, lo avete svuotato delle sue prerogative. State tradendo tutti i principali dettati dei nostri Padri costituenti, ma quel che è peggio, in questo momento di difficoltà, è che state tradendo la fiducia del Paese. Il vostro è un tradimento delle categorie più indifese: i lavoratori precari e senza tutele, le famiglie che vedono sempre più perdere il proprio potere d'acquisto e non arrivano a fine mese, le donne a cui volete concedere solo una parità di facciata e far cassa dalle loro pensioni, il Sud, che sta vivendo una crisi senza pari e che di nuovo vede andar via le sue menti più brillanti, i giovani della potenziale classe dirigente meridionale.

Poi ho dovuto rassegnarmi. Evidentemente, nonostante i tanti voti raccolti da questa maggioranza nel Mezzogiorno, Governo e Ministro dell'economia e delle finanze avevano pensato di dover rivolgere l'attenzione soltanto alle aree più forti del Nord del Paese. Oggi, una settimana dopo la presentazione del DPEF presso la Commissione bilancio del Senato, la scena è completamente cambiata. Il Presidente del Consiglio annuncia un piano speciale per il Sud: i mitici fondi FAS di un tempo, poi ampiamente utilizzati e svuotati a mo' di Bancomat per le spese quotidiane del Governo, si annuncia che saranno magicamente nuovamente resi disponibili per le aree deboli; e non finisce qui. A favore della spesa per il Sud si parla di una nuova Agenzia centrale, sul modello della Cassa, e financo di un Ministero appositamente dedicato. C'è da non credere ai propri occhi! Dopo un lungo tempo di rimozione o al massimo di citazione dei vizi pubblici di un Sud sempre e solo spendaccione, accattone, e chi più ne ha più ne metta, oggi d'improvviso l'antica questione meridionale sembra tornata al centro, quanto meno dei titoli di prima pagina. Per guardare all'Italia rovesciata, per all'Italia rovesciata, per l'allargamento dei cordoni della spesa è bastato alla maggioranza l'annuncio di un nuovo partito del Sud. Si potrebbero fare considerazioni squisitamente politiche in proposito, ma per la verità vorrei guardare un po' di più alla società. Tra l'altro, insieme alla stravaganza della derubricazione del Mezzogiorno dal DPEF, va richiamata un'altra questione altrettanto delicata: il giudizio sulla crisi. L'impressione, ampiamente confermata dagli interventi pubblici e parlamentari del ministro Tremonti, è quella di una minimizzazione degli impatti della crisi globale nel nostro Paese, che viene sempre descritta con accenti edulcorati ed effetti sottovalutati, sia per il presente che per la prospettiva, come a dire che non è cambiato molto e soprattutto che non dovrà cambiare molto del nostro modello di sviluppo. Molte parole sono state spese per rassicurare ed infondere fiducia contro i catastrofisti, che non vedrebbero gli eccellenti risultati dell'azione di governo e la tenuta sociale e produttiva dell'Italia nell'Unione europea. Per finire, con l'annuncio di ieri secondo cui saremmo già al *day after* e non sarebbe successo nulla. Peccato, però, che il problema non sia di pura comunicazione politica e che per dare voce alla realtà non servano

Nella mia Regione ogni giorno scompaiono centinaia di posti di lavoro e solo per i più "fortunati" c'è il ricorso agli ammortizzatori sociali. Sono circa 53.000 nel 2009 - solo nel 2009 - i lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria. si parla della Campania, non dell'Emilia-Romagna: una regione in cui se ad una famiglia viene meno un reddito viene meno il reddito per la famiglia stessa perché, come è noto, da noi solo una donna su quattro lavora fuori casa. E sempre in materia di occupazione femminile, un tema che si presta particolarmente ai buoni propositi e alle pessime pratiche, vorrei sottolineare che nelle otto Regioni meridionali, per effetto dei tagli deliberati dal Governo sulla scuola che, come si sa, è un comparto di lavoro femminile, salteranno 20.000 cattedre e tra queste i pensionamenti sono poco più di 13.000. Del resto - lo voglio dire chiaro e forte - la scuola campana è la più colpita dai tagli del Governo.

Seguono la Sicilia, con 5000 posti tagliati, la Puglia con 3.600 e la Calabria con 2.800. È inutile dire - e non voglio annoiare con i numeri dei tagli al Nord e al Sud - che sono stati usati pesi e misure diverse, a tutto svantaggio del Mezzogiorno. Queste sono solo alcune delle questioni che emergono a proposito della crisi del mercato del lavoro, in questo caso grazie alle politiche dirette del Governo. Poi ci sono quelle che non si vedono, ma si conoscono fin troppo bene, e cioè, nel Mezzogiorno, il conseguente, ulteriore allargamento dell'area del lavoro e dell'economia sommersa, con tutti gli effetti di maggiore degrado e impoverimento del nostro apparato produttivo, a cominciare da quelli del riciclaggio, portati all'attenzione della Commissione antimafia dal governatore Draghi. L'approccio del DPEF e il punto di vista che ci ha rappresentato il Ministro intervenendo alla Commissione bilancio sembrerebbero voler essere quelli del buon padre di famiglia, che a fronte di una temperie esterna di proporzione inaudita sceglie per prudenza un comportamento, vorrei dire, zen: agire il meno possibile per ridurre i danni. Si tratta di un approccio che non regge alla prova dei fatti, della crisi e dei dati di cui disponiamo; dati che ci parlano di una disoccupazione al 9 per cento, di un vero e proprio collasso del PIL (-5 per cento); dati che danno conto di una pesante stagnazione aggravata da una drammatica crisi della finanza pubblica, e infatti aumentano spesa, debito, spesa corrente e, incredibilmente, aumenta di tre punti anche la pressione fiscale, a fronte di una sensibile riduzione del gettito. Dunque, dopo un anno di autosufficienza, il buon padre di famiglia non è tale se continua a ripetere che tutto va bene e a rinunciare a cambiare. Non è vero che va bene, non è così e tra l'altro sono stati commessi errori che dovrebbero essere riconosciuti, per esempio tutti quelli legati all'avvio della legislatura, quando ingenti risorse sono state impegnate per azzerare l'ICI sulla prima casa, privando i Comuni di risorse proprie, in gran parte non ancora restituite, che avrebbero potuto, diversamente, essere investite con priorità per quelle misure anticicliche di sostegno della domanda interna, così come proposto dal Gruppo del Partito Democratico. Noi abbiamo fatto molte proposte, e tutte proposte serie; quando ci avete risposto - e non sempre ci avete risposto - avete sostenuto che non era nelle possibilità e nell'interesse dell'Italia promuovere politiche anticicliche che avrebbero avuto effetti sul *deficit*, che a differenza di altri Paesi dell'Unione noi non possiamo permetterci. Ora, i dati mettono in luce che la vostra posizione rinunciataria non è sostenibile, in nome della tenuta sociale, ma anche della tenuta contabile del Paese, e che avete commesso un grave errore di autosufficienza autosufficienza nel rifiutare di aprirvi all'apporto delle proposte dell'opposizione, che invece si è dimostrato valido e lungimirante. È chiaro infatti nel DPEF che, nonostante il Governo agisca sulla proposta di bilancio per dare messaggi rassicuranti, sul fronte sulla spesa alcune voci continuano ad essere fuori controllo alimentando la crescita del debito pubblico. Sarebbe semplicemente onesto prendere atto che l'economia italiana va male e peggio di quasi tutti i Paesi dell'Unione, che la finanza pubblica è in crisi grave, che tutto ciò avviene, a differenza di tutti gli altri Paesi europei, senza che il Governo abbia voluto assumere misure di contrasto, che c'è un peggioramento dei saldi di bilancio e che questo accade anche per un aumento dell'evasione fiscale che aggrava la caduta del gettito e infine che, nonostante i tagli tanto gravi, la spesa sembra crescere oltre le previsioni e senza controllo. Ecco perché è assolutamente necessario sottoporre ad una profonda revisione le politiche di sviluppo del Governo e abbiamo il dovere, come Paese, di scommettere sulle possibilità che questo periodo di crisi tanto grave e intenso serva per progettare un futuro diverso, affinché proprio il carattere tanto radicale della crisi, certo internazionale, possa essere utilizzato per cambiare alcuni caratteri di fondo e di funzionamento della nostra società. Questo sarebbe quanto mai auspicabile per tutta l'Italia e per il nostro Mezzogiorno in particolare. Io che mi considero una migrante a Napoli, in mezzo a tanti dubbi, a tante delusioni per tanti progetti di cambiamento che abbiamo iniziato in questi anni e poi bruscamente interrotti, mi sono fatta modestamente l'idea che quello che più è mancato in questi anni al Mezzogiorno è stata la continuità di politiche riformatrici nazionali valide per tutto il Paese, politiche che richiedono agende largamente condivise, respiro largo e tempi lunghi. Oggi certamente un banco di prova per riprendere un cammino di riforma è rappresentato dai decreti legislativi sul federalismo fiscale, ma certamente una priorità assoluta per il Mezzogiorno è una moderna politica di inclusione, di lotta alla povertà e di cittadinanza, accompagnata da una vera e propria esplosione di imprenditorialità in settori strategici tali da valorizzare risorse, vocazioni e meriti. Per concludere, ieri sera Mediaset ha mandato in onda un bellissimo film, che forse molti avranno visto, "L'illusionista". Ecco, ho pensato, forse questo film sarà piaciuto molto anche al ministro Tremonti, ma sicuramente questo modo di procedere

Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatori, nell'esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 è necessario far riferimento, seppur per larghe linee, al quadro economico in cui si inserisce, in quanto documento tecnico di strategia politica che rivela le aree socio-economiche sulle quali si concentrano l'attività legislativa e gli interventi dell'Esecutivo. I rischi per l'economia mondiale provengono in primo luogo dall'incertezza ancora presente nel sistema finanziario internazionale. In Italia, in modo particolare, permane l'esigenza di garantire la normalità dell'erogazione dei flussi di credito. Il peso delle imprese manifatturiere nel nostro Paese richiede, infatti, linee di credito agili per non intaccare i livelli occupazionali. Secondo recenti stime sono a rischio, entro la fine dell'anno, tra i 500.000 e gli 800.000 posti di lavoro.

un retroeffetto negativo. Tuttavia, il rischio che comporta un simile atteggiamento sta nel ritardo della ripresa economica, che deve essere scongiurato. Il nostro Paese deve marciare alla stessa velocità delle economie più sviluppate. I finanzieri hanno l'obbligo, dunque, di avere occhi aperti anche per chi ha perso o potrebbe perdere il proprio lavoro e di sostenere,

provengano dal Governo esortazioni e interventi concreti per indurre le banche ad una maggiore fiducia. Le banche italiane hanno utilizzato soltanto una piccola parte dei 12 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo per fronteggiare il *credit crunch*. Contemporaneamente, come si evidenzia nella relazione allegata al DPEF, l'intervento statale a sostegno delle imprese è stato nel 2008 considerevole: anche qui circa 12 miliardi di euro, di cui quasi la metà già effettivamente erogati. Sappiamo tutti leggere ed interpretare i dati del DPEF. La ripresa del prossimo anno (+ 0,5) significa ancora livelli di PIL inferiori a quelli di due anni fa. Dovremo perciò attendere altri due anni per recuperare il terreno perduto in termini di ricchezza prodotta rispetto al 2008. Potrebbe andare meglio per il tasso di disoccupazione, che si attesterà

resta quella del lavoro. Dobbiamo riconoscere al Governo un grande impegno nei vari provvedimenti anticrisi adottati: circa il 22 per cento delle risorse stanziate per il 2009, nonché il 46 per cento di quelle disposte per il 2010

tra il primo semestre 2009 e quello dell'anno scorso ha fatto un balzo di oltre il 280 per cento, soprattutto nei settori meccanico, metallurgico e chimico. Questa crisi si supererà solo sostenendo la domanda reale e se le aziende riprenderanno ad investire; riguardo al settore degli ammortizzatori sociali, forse occorrerà riconsiderare anche la misura della cassa integrazione. Mi pare positivo, sempre in sempre in termini di attenzione al lavoro, l'impegno del Governo a mantenere la sostenibilità del sistema del Welfare e delle politiche giovanili, anche attraverso un più efficiente raccordo tra scuola e mercato del lavoro e il rilancio del contratto di apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mondo del lavoro. Il Documento ricorda inoltre che è in fase di avvio un piano di azione sull'occupazione femminile, incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro, sulle norme che favoriscono la diffusione del lavoro a tempo parziale, su misure di incentivazione per l'assunzione delle donne con i contratti di inserimento al lavoro nelle aree svantaggiate e sulla sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e di assistenza alla persona. Qualcosa per il Sud c'è, piccolo piccolo. il Sud c'è, piccolo piccolo. Ci sarebbero ancora tante altre cose da aggiungere. Il Documento è pregno di sostanze interessanti ed importanti per il futuro del nostro Paese, come per esempio l'impatto del nuovo indice di calcolo per gli incrementi salariali, stabilito nell'accordo del gennaio scorso con i sindacati,

Esso, infatti, si configura come un mero catalogo di impegni, privo di ogni garanzia sulla certezza dei finanziamenti e soprattutto sui tempi di avanzamento delle opere. Su 10.138 milioni di euro di risorse pubbliche stanziate dal CIPE per le infrastrutture nella delibera del 6 marzo scorso, poi articolate per singoli interventi dallo stesso Comitato nella seduta 26 giugno, solo 83,4 milioni saranno spesi effettivamente nel corso del 2009, mentre 2.441 milioni, pari al 24 per cento troveranno spazio nel biennio 2009-2010. Sono dati importanti. Il grosso della fetta, però, produrrà pagamenti solo successivamente, cioè nel 2011 per 3.612 milioni e dal 2012 in poi per 4.091 milioni di euro, ovvero il 40 per cento dell'intero ammontare deliberato. Ciò significa una cosa fondamentale, cioè che questo Governo ha deciso di risolvere la grave crisi infrastrutturale rinviando di anno in anno l'erogazione dei finanziamenti. Questo purtroppo equivale, cari colleghi, equivale, cari colleghi, a decidere di non decidere se e quando asseverare il definitivo completamento delle opere già cantierate. Gli 800 milioni di euro stanziati per il Mose di Venezia, ad esempio, saranno spesi solo per un decimo quest'anno (80 milioni di euro), nonostante l'opera sia in piena realizzazione. Avremo poi 320 milioni nel 2010, 240 nel 2011 e 160 dal 2012. Anche per quanto riguarda l'Italia meridionale, nonostante si ribadisca l'impegno al completamento della Salerno-Reggio Calabria e venga sottolineata l'importanza strategica dell'asse ferroviario Napoli-Bari, della statale 106 Ionica, nonché degli *hub* portuali e interportuali di Augusta, Brindisi e Taranto, la tempistica con la quale i finanziamenti potranno essere di fatto erogati appare completamente insostenibile e contraddittoria. Con riferimento, ad esempio, al completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria (macrolotto 3, parte 4) si rileva che nonostante per tale intervento sia stato autorizzato un finanziamento per 345 milioni di euro, 205 di questi potranno essere assegnati solo dopo il 2011. Preoccupa, inoltre, l'incertezza dei dati relativi ai tempi di progettazione e di realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 di Milano, quali le linee metropolitane M4 ed M5, come pure i dati per attivare gli assi infrastrutturali strategici all'interno del Corridoio 5 Lisbona-Kiev, il traforo del Frejus, il traforo del Brennero (Corridoio n. 1), il terzo valico tra Milano e Genova e il completamento della TAV fino a Venezia.

in che modo questa operazione potrà partire, perché, al di là del fatto che il tema è stato inserito nell'agenda politica da Matteoli, pare non esserci altro. Nell'Allegato infrastrutture, infatti, si parla sì di Alta velocità ma per quanto riguarda l'asse Milano-Verona e, in particolare, per la tratta Brescia-Treviglio. La priorità, e relativi finanziamenti, sono dunque legati alla tratta Brescia-Treviglio. Si parla anche della Verona-Venezia, ma la sua realizzazione rimane condizionata alla soluzione del nodo di Vicenza. Infine, si fa presente che: «in realtà si sta cercando di dare attuazione all'intero asse ferroviario Torino-Trieste». Insomma, le intenzioni, mi pare di averle già elencate, forse ci sono, ma i problemi da affrontare sembrano essere enormi per non parlare delle risorse, sempre più ingenti, sia per quanto riguarda la Verona-Venezia sia per la Venezia-Trieste. appare inammissibile la decisione di questo Governo di destinare 1,3 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e 904 milioni di euro di euro per gli interventi a terra connessi alla realizzazione del ponte sullo Stretto, quando le stesse risorse potrebbero essere davvero utilizzate, ad esempio, per affrontare l'emergenza del terremoto avvenuto il 6 aprile scorso in Abruzzo, o per adeguare la viabilità stradale in Sicilia e Calabria. Infine, per quanto riguarda il progetto di ampliamento della banda larga, altro tema molto importante, si considerano spropositate le stime su ipotesi di investimento di 1,471 miliardi di euro per lo sviluppo di reti telematiche di nuova generazione, dal momento che un iniziale finanziamento, stimato in circa 800 milioni, sarà nella realtà inferiore alla previsione iniziale. Per tali ragioni, onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori presenterà una risoluzione per impegnare il Governo su cinque punti: in primo luogo, a porre in essere un'efficace selezione delle priorità, una pianificazione finanziaria da elaborare e aggiornare in funzione delle reali necessità del Paese, assicurando un percorso di crescita delle risorse pubbliche ed indicando in modo certo, trasparente e puntuale

pari a 1,3 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e 904 milioni di euro per gli interventi a terra. In a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato sia ad incrementare, sia ad accelerare l'erogazione delle risorse volte a garantire l'avanzamento dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dell'asse ferroviario Napoli-Bari, della statale 106 Ionica, nonché degli *hub* portuali ed interportuali individuati dall'allegato infrastrutture. a velocizzare i tempi di progettazione e di realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 di Milano, quali le linee metropolitane M4 e M5, come pure i dati per attivare gli assi infrastrutturali strategici all'interno del corridoio n. 5 (Lisbona-Kiev), traforo del Frejus, traforo del Brennero, il terzo valico della Milano-Genova ed il completamento dell'Alta velocità fino a Venezia. Per ultimo, si chiede al Governo di destinare adeguate risorse per garantire la piena attuazione del progetto di ampliamento della banda larga, mantenendo fermo l'iniziale finanziamento di 800 milioni di euro destinati a tal fine.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, come sappiamo, questo sarà l'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria; dal prossimo anno lo sostituirà, se sarà approvata la nuova legge di finanza pubblica, già licenziata dal Senato in prima lettura, il DPF (Decisione di finanza pubblica). Forse per questo motivo, il Ministro ed il Governo si sono ingegnati a fare in modo che nessuno ne rimpiangerà la portata: un Documento previsionale piatto, reticente quanto a informazioni sui livelli e sulla composizione delle entrate e delle spese, in cui si certifica, se consideriamo i saldi netti, che non ci sarà alcuna manovra per rilanciare i conti pubblici nel 2010, e che si resta, come siamo stati per tutto il corrente anno, in linea di galleggiamento, aspettando e sperando nell'evoluzione degli sviluppi futuri. Insomma, se stiamo al DPEF e al Governo, ci dovremmo limitare a fidarci: lasciarci cullare nelle braccia del Ministro dell'economia, che tutto prevede e che, per il potere che ha concentrato su di sé in quest'anno, approfittando della crisi, tutto dispone. Ma come si fa a fidarsi? È lo stesso DPEF, pur così smilzo ed autocelebrativo, a certificare, con dati forniti dal Governo, che l'economia italiana sta conoscendo una *performance* peggiore di quasi tutti i Paesi europei; che la finanza pubblica è ripiombata in una crisi gravissima, tanto che dopo 18 anni si torna a generare un disavanzo primario; che ciò avviene senza che il Governo (unico in Europa) abbia assunto misure discrezionali per contrastare la crisi. Infatti, al di là delle cifre roboanti con cui si è scimmiottato il gioco delle tre carte negli ultimi mesi, l'entità netta degli interventi a sostegno dell'economia, messi sin qui in atto dal Governo, è stata di circa 3 miliardi: davvero pochissimo se rapportato alla gravità e ai costi sociali della crisi. Inoltre, il Documento certifica che, nonostante i tagli introdotti, la spesa pubblica cresce ben oltre le previsioni e senza controlli. Infine, assistiamo a un peggioramento dei saldi di bilancio, che deriva anche da un aumento dell'evasione fiscale, che accentua la caduta del gettito e delle entrate complessive. Su quest'ultimo aspetto i nodi stanno venendo al pettine. Il crollo delle entrate, pur così rilevante, e che si vuole far dipendere dalla mera conseguenza del calo previsto del PIL cento), non tiene in realtà conto né dell'incidenza dovuta alla ripresa dell'evasione, né delle sue probabili dinamiche ulteriormente incrementali, con particolare riferimento alle imposte indirette. In questi mesi si sono a più riprese sottolineati i buoni risultati relativi all'accertamento e alla riscossione. Il fatto che gli accertamenti siano arrivati a 20 miliardi e che la riscossione raggiunga i 2 miliardi è un dato positivo, frutto di un aumento dell'attività di contrasto, dell'affinamento delle banche dati fruibili, di un'efficienza operativa che va a merito di un investimento politico non solo dell'oggi, e soprattutto delle capacità e impegno delle Agenzie fiscali e della Guardia di Finanza. tali sforzi, importanti e apprezzabili, rischiano di venire vanificati, se non si riduce la propensione dei contribuenti a evadere a monte; propensione che purtroppo i dati sull'IVA sembrerebbero dimostrare essere nettamente in aumento. Forse su questo punto il DPEF, anziché sorvolare, avrebbe fatto bene a soffermarsi. Ce lo suggeriva anche il governatore Draghi, interrogandosi su come interpretare il divario tra la dinamica del gettito dell'IVA (in riduzione nel 2008) con quella della base imponibile del tributo stesso che invece, per converso, è in aumento, seppur lieve. Non è questo un indicatore inquietante di un possibile crescere dell'evasione? Forse è la cartina di tornasole che il vostro tentativo di conciliare la netta inversione di rotta rispetto all'azione intrapresa dal Governo nella precedente legislatura in tema di evasione, salvaguardando comunque il gettito fiscale, con lo spostamento dell'attenzione dai piccoli e medi (lavoratori autonomi e piccole-medie imprese) ai grandi contribuenti (persone fisiche con indici elevati di capacità contributiva e grandi imprese) e quindi la modifica di atteggiamento e di focalizzazione e di attenzione, in realtà non può funzionare. Così come è indubbio che l'abbassamento consistente delle sanzioni, non compensato da un aumento della probabilità di essere scoperti, unito ad una situazione di crisi economica caratterizzata da difficoltà di accesso al credito specie per i piccoli e medi operatori, aumenta la convenienza e la tentazione di evadere. Il rischio della strategia che avete messa a punto è che l'adempimento spontaneo sia disincentivato, anche perché si può pensare che, se scoperti, si potrà definire il debito di imposta con sanzioni agevolate. Insomma, aver abolito le limitazioni nell'uso di contanti e di assegni, la tracciabilità dei pagamenti e la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati, insieme a numerosi altri adempimenti per il controllo e la trasparenza, come il ridimensionamento della solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore, può aver rafforzato - non lo nego - qualche simpatia di breve momento verso la maggioranza tra l'elettorato delle piccole partite IVA, per l'effetto psicologico di sentirsi meno stretti da vincoli e incombenze. Ma, alla prova dei fatti, voi, e anche loro, che per la grandissima parte sono contribuenti responsabili, dovreste prendere atto che i danni prodotti sono ben superiori, e porvi rimedio: ma temo che questo, purtroppo, ci si guarderà bene dal farlo. E così, le conseguenze sono quelle inevitabili: una pressione fiscale che tocca il 43,4 per cento del PIL nel 2009 e rimane su livelli prossimi al 43 per cento per tutto il periodo di previsione del DPEF, fino al 2013. Valori che ci collocano ampiamente sopra la media degli altri Paesi dell'area euro e che sono attestati sul nostro massimo storico. Capisco che avvertiate un certo imbarazzo e persino un po' di senso di colpa, per l'abisso che c'è tra quello che avete sbandierato e propagandato agli italiani negli anni passati e quello che in concreto state facendo ora che siete al Governo: evitate però la meschinità come avete fatto la settimana scorsa in quest'Aula, come esimente una sorta di peccato originale che sarebbe da ricondurre alle politiche economiche e fiscali attuate nei due anni di governo del centrosinistra! Noi i conti, compresi quelli del contrasto all'evasione ed all'elusione, ve li abbiamo lasciati in ordine: lo ha certificato l'Europa e ce l'ha riconosciuto il vostro DPEF l'anno scorso. La responsabilità di questa situazione è tutta e solo vostra: voi avete allentato il contrasto all'economia irregolare e, conseguentemente, determinato le condizioni perché ci sia un aggravamento del peso sui contribuenti ligi al dovere fiscale, soprattutto tra i lavoratori dipendenti e i pensionati e per per quelle imprese che agiscono correttamente e subiscono una concorrenza sleale. Certo, il DPEF, a parole, attribuisce grande importanza alla lotta all'evasione. Peccato non ci dica nulla su come invertire la tendenza in atto e dar seguito all'intento. Il ministro Tremonti confida molto nel federalismo fiscale. È legittimo attendersi dei ritorni positivi, ma quel traguardo è lontano anni e poi l'ambito della possibilità di svelare omissioni è necessariamente circoscritto. Le indagini dagli esiti più promettenti restano quelle da svolgere sulle imprese e qui il ruolo fondamentale è quello delle Agenzie delle entrate e della Guardia di finanza, che fanno cose egregie ma potrebbero incidere maggiormente con il supporto di quelle misure subito cancellate Così, poiché la criticità dei conti pubblici preme e le necessità di cassa incombono, ecco pronta dietro l'angolo - la approveremo alla fine di questa settimana - una terza edizione dello scudo fiscale per il rientro dei capitali all'estero. Ne parleremo quando approveremo quel provvedimento, ma devo dire che questa è una mortificazione odiosa per i contribuenti che sopportano il carico di quel 43,4 per cento di pressione fiscale

bisogna perseguire l'obiettivo di stabilità della normativa in materia di accertamento e soprattutto consolidare una cultura di non tolleranza dell'evasione. Ebbene, fate e farete esattamente il contrario e questo credo sia discutibile e certamente discutibile e certamente censurabile, e soprattutto che penalizzi i corretti contribuenti, i quali avrebbero bisogno di sentire lo Stato molto più dalla loro parte e non dalla parte di coloro che portano i capitali all'estero e poi vengono assolti per un piatto di lenticchie!

economico-finanziaria, e soprattutto tutte le considerazioni, mi sono sentito finalmente soddisfatto perché, contrariamente a quanto ha detto il collega che mi ha preceduto, dopo 15 legislature vedo finalmente realizzato qualcosa di di concreto in un momento difficilissimo perché, come abbiamo detto, oltre che la crisi internazionale affrontiamo anche alcuni danni fatti in due anni dal Governo precedente. Il problema, però, è subito sorto nell'immediato quando, da buon parlamentare eletto in Sardegna, sono andato a controllare le risorse. Quindi, pur sapendo che le risorse sono estremamente ridotte e che devono essere naturalmente investite uso questo termine per cercare di rilanciare la nostra Nazione - vado a leggere, per esempio, per le infrastrutture essenziali e fondamentali per la Nazione, quanto destinato per la mia Sardegna: 18 milioni

che sta tanto a cuore al Presidente; una Regione che insieme alla Sardegna è l'unica regione insulare e le posso confrontare perché hanno la stessa estensione. Una ha la fortuna di essere ad un tiro di schioppo dal continente e l'altra è molto più lontana;

pari a 5.495.000.000. Vuol dire che la Sicilia, che sicuramente ha bisogno di queste risorse, riceverà

se prima i parlamentari rappresentavano la Nazione e dovevano soprattutto interessarsi alla Nazione, oggi per una scelta condivisa, *bipartisan*, di trasformazione di uno Stato sempre più in senso federalista, voi dovete - come sto facendo io - sempre più avvertire ciò che abbiamo avvertito in questi giorni: i parlamentari eletti in una regione dovranno giustamente difendere quanto più possibile gli interessi della propria regione. Quindi sono qui presente - ed ho voluto prendere la parola - anche se solo per cinque minuti, parlando a braccio e non leggendo alcunché, per chiedere al Governo di riequilibrare e di rendere tollerabile ed equilibrata una destinazione di risorse, perché è giusto che ci siano dei parametri

voluto immediatamente, nella sua risoluzione, porre il problema della Sardegna, che era la Regione che più pagava questa disuguaglianza che ritengo umiliante, perché i parlamentari come me sono sempre stati ligi al mandato ricevuto dai propri elettori e

capite che oggi, per la situazione che stiamo vivendo, una Regione come la mia, che sta vivendo una situazione drammatica, che stranamente vive più del Nord la crisi (mentre in passato erano le Regioni del Nord che subivano maggiormente il problema) non può affrontare questa disuguaglianza. perché, in conclusione, rivolgo un appello al vice ministro Vegas, che so essere stato sempre molto attento al giusto equilibrio nella distribuzione tra le Regioni, e soprattutto alla sensibilità non solo del Governo ma di questa maggioranza, perché al più presto, nei prossimi provvedimenti e nel bilancio, venga riequilibrata la destinazione delle risorse, per non creare questa ingiustizia che sarebbe intollerabile e ci porterebbe a degli atti che non fanno parte della nostra cultura.

mi sembra che in questo dibattito finora non sia stato affrontato come dovuto un tema peraltro fondamentale per la manovra di finanza pubblica

che il Patto di stabilità interno sta producendo sul sistema degli enti locali italiano. Da un recente documento che mi è stato fornito dal Consiglio nazionale dell'ANCI risulta che circa il 43 per cento degli investimenti pubblici è stato realizzato dai Comuni, che a tal fine hanno impegnato oltre un quarto delle loro risorse disponibili. sono note le proteste, ormai unanimi, di tutte le associazioni imprenditoriali, dai costruttori alla Confindustria, agli artigiani, alle cooperative, i quali giustamente lamentano il fatto che, non potendo i Comuni pagare neanche gli stati di avanzamento dei lavori appaltati, tutto questo, proprio a causa di quei nefasti vincoli del Patto di stabilità interno, produce una situazione di allarme gravissimo per la crisi, e molte di queste aziende rischiano addirittura in termini di fallimento. Nel decreto anticrisi che esamineremo nel corso dei prossimi giorni - ritengo senza molti margini per cambiarlo - la maggioranza la maggioranza ha proposto alla Camera un emendamento che è stato ritenuto di sollievo per i Comuni e che aumenta l'ammontare dei residui passivi in conto capitale che si possono utilizzare. Ancora una volta l'ANCI valuta che questo emendamento valga circa 800-1.000 milioni di euro. Ma c'è un altro numero che preoccupa davvero e rispetto al quale questa è davvero una goccia nel mare e cioè la manovra economica triennale, che questo DPEF conferma, la quale prevede che a legislazione vigente, nel triennio 2009-2011, i Comuni debbano migliorare i propri conti di più di 4,3 miliardi di euro, che si traducono in una riduzione del 18 per cento della spesa totale. Mi rivolgo, oltre che al vice ministro Vegas, al presidente Azzollini, che vedo in Aula, ed al collega Garavaglia, relatore del DPEF, che sappiamo essere sensibile a questi temi. È assolutamente indispensabile che il Parlamento metta mano a questa situazione, che si sta davvero traducendo in un aggravio pesantissimo per le famiglie e le imprese, in un momento in cui i Comuni dovrebbero essere invece messi in condizione di porre in essere una manovra anticiclica, quindi di sostenere l'economia e di non deprimerla. che è probabile vi sia un'abolizione delle sanzioni per quelle amministrazioni locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2009. Anche noi quando discutemmo del federalismo fiscale sostenemmo che, in assenza di altre misure, questo comunque poteva essere un provvedimento da prendere, ma non è serio che si proceda in questo modo. Fra l'altro, e concludo, nell'esame del provvedimento sul federalismo fiscale e nell'introduzione in questo di norme importanti come il patto di stabilità ed il patto di convergenza, abbiamo verificato l'accordo tra le diverse parti politiche sulla necessità di dare luogo ad una differente procedura di costruzione di questi meccanismi, che sia partecipata partecipata e che veda pertanto effettivamente il sistema delle Regioni e delle autonomie locali in condizione di contribuire fattivamente a definire obiettivi che poi si impegnano a rispettare. Per questo, mi rivolgo sia al relatore, senatore Garavaglia, che al vice ministro Vegas affinché sia data soluzione a tale problema. Ritengo in particolare che, fino a quando ciò non sarà fatto, ci troveremo di fronte ad una situazione che, indipendentemente dalle parti politiche, sarà necessario affrontare. Responsabilità vorrebbe che lo si facesse subito, a partire dalla risoluzione di approvazione del presente

*(PD)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 non contiene previsioni programmatiche significative per il settore agroalimentare. Il contributo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali introduce misure che, lungi dal ristabilire l'operatività del sistema, rispondono esclusivamente ad una logica di ordinaria amministrazione

appare quale mera misura compensativa rispetto ai tagli operati dal Governo sia con il decreto-legge n. 112 del 2008 sia con la legge finanziaria per La realizzazione delle misure e degli interventi per il settore, secondo quanto indicato nelle premesse dell'Allegato n. 3 al Documento LVII, n. 2, sarà funzionale all'andamento dell'economia e al rispetto dei criteri di rigore nella gestione del bilancio pubblico. Viene completamente ignorata la questione dell'indebitamento delle aziende agricole; non è affrontato il problema del credito d'imposta; non viene fatta menzione di misure innovative per l'accesso al credito; l'internazionalizzazione delle imprese viene affidata alla previsione di uno stanziamento di soli 20 milioni di euro. Il Documento LVII, n. 2, e i suoi allegati ignorano il settore della pesca che ha contribuito e contribuisce ancora alla prosperità e alla crescita economica del Paese. In definitiva, non è quindi possibile parlare di politiche di rilancio del settore agroalimentare all'interno del DPEF approvato dal Governo. Tutto ciò accade all'interno di una fase molto delicata che vede le imprese agricole e alimentari sottoposte, al pari di ciò che sta accadendo al sistema economico nazionale, in modo diretto e indiretto alle gravissime conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale, i cui segnali sono ben manifesti:

i redditi degli agricoltori sono ovunque in calo e le aziende agricole sono sempre più indebitate; difficoltà crescenti per gli agricoltori si stanno verificando nell'accesso al credito; le imprese agricole sono assoggettate a tassi di interesse più elevati rispetto a quelli praticati dal sistema bancario ad altri settori produttivi. È dunque ben giustificato il pessimismo diffuso anche tra gli operatori dell'industria alimentare, come dimostrano le indagini periodiche condotte dall'ISMEA nell'ultimo anno. La crisi internazionale in atto ha avuto ripercussioni sull'intero sistema agricolo europeo e i principali Paesi dell'Unione hanno adottato manovre anticrisi includendo misure specifiche per il rilancio competitivo del comparto come accaduto in Francia, dove il ministro dell'agricoltura Barnier ha ha varato un piano di 250 milioni di euro per sostenere i redditi degli agricoltori. Il Gruppo del Partito Democratico ha insistito qui, al Senato, fin dai primi mesi di quest'anno sulla necessità di adottare interventi immediati ed organici a sostegno del comparto. Lo ha fatto in particolare attraverso la presentazione di una mozione, a prima firma della collega senatrice Pignedoli, Capogruppo in Commissione agricoltura. Manca il tempo, signor Presidente (vado a concludere il mio intervento), per ricordare i punti salienti che caratterizzano quella nostra iniziativa e dunque non do lettura di quanto ho di seguito indicato,

di indebitamento. In mancanza di precise indicazioni in grado di offrire prospettive concrete al comparto agroalimentare, questo DPEF - che presenta innumerevoli carenze sul piano della sua impostazione generale e nei singoli settori d'intervento - non può trovare alcun avallo da parte del Partito Democratico. **Testo

alcune necessarie riflessioni sui primi 14 mesi del Governo Berlusconi, prima ancora di passare alla valutazione sulla programmazione economica e finanziaria in esso contenuta:

perché ha permesso di mantenere la coesione sociale, tranquillizzando le famiglie che al risparmio danno un particolare valore, specialmente perché è frutto dei loro sacrifici e rappresenta l'unica fonte di sicurezza

da parte dei privati nelle casse dello Stato. Vorrei richiamare qui anche il Trattato di amicizia con la Libia, che ha chiuso una pagina di storia, un periodo di risentimenti e di rivendicazioni, aprendone uno nuovo di collaborazione e pacificazione. Esso comporta anche 180 milioni di euro all'anno di investimenti ad esclusivo vantaggio delle imprese italiane: si tratta quindi di un altro sbocco eccezionale per l'economia in un momento di sofferenza.

con 4.700 gru, con 3.500 edifici che devono sorgere, con case in costruzione, grattacieli da sogno destinati a modificare l'assetto urbano, metrò in arrivo per garantire infrastrutture all'altezza della grande sfida dell'Expo, nuove strade e tunnel per velocizzare il traffico. Tutto questo mi riempie di orgoglio perché la mia identità

che procedono in parallelo, per un totale di 15 miliardi di euro fino al 2013 e ai primi mesi del 2014, con un cronoprogramma che nel corso dell'audizione del vice ministro Castelli abbiamo avuto l'opportunità di vagliare per singola infrastruttura,

quelli reali a quelli ambientali. In un simile contesto avere la forza di reagire e di dare impulsi positivi all'economia diventa il messaggio principale che può venire dalla classe politica ed il Governo

dolci parole, che si ascoltano con piacere, specialmente quando poi, guardando anche al completamento del capitolo, si afferma che in assenza di un'operazione incisiva capace di diventare reale in un arco temporale certo si rischia di rendere irreversibile lo stato di arretratezza del Sud. Pertanto, quando il nostro Presidente del Consiglio parla di un piano innovativo per il rilancio del Sud noi confermiamo la nostra fiducia nella sua capacità di sintesi e nella sua politica nazionale. Il PdL è un partito nazionale. Il Sud è una questione nazionale; quindi, va impostata e affrontata con una politica nazionale. Vorrei concludere il mio intervento rifacendomi all'invito del presidente Ciampi che ha dato impulso a tutti noi, ha scosso la nostra sensibilità e ha richiamato il nostro senso di responsabilità per guardare ad un'Italia che deve crescere e che può crescere solo nell'unità d'intenti. Cerchiamo di fare, maggioranza e opposizione, una politica corretta, svolgendo il confronto in termini

I ministri Gelmini e Bondi, dopo i pesanti tagli dello scorso anno, avevano dato a questo appuntamento l'idea di un primo ravvedimento nel ripristino di alcune risorse fondamentali. Nell'ultima audizione in Commissione il ministro Gelmini aveva affermato, ribadendo il concetto due volte, che nel primo anno di attuazione della riforma erano stati risparmiati 2 miliardi di euro a fronte dei 600 miliardi di euro previsti e che sarebbero stati reinvestiti nel merito degli insegnanti migliori,

Il Ministro si consola dicendo che si è ottenuto una scuola più severa che boccia di più. Siamo sicuri che questo è un segnale di ottimismo, di miglioramento,

ha detto che il fallimento, se si vuole la sconfitta finale, non è dei ragazzi bocciati ma della scuola intesa come sistema formativo ed educativo nel suo insieme. Credo che non dovrebbe succedere che solo alla fine della fase fondamentale del cammino scolastico ci si renda conto che uno studente non è idoneo a proseguire o ad accedere ad una professione. Penso sia un segnale preoccupante che può indicare che la nostra scuola non è in grado di capire ed interessare i nostri ragazzi e deve ricorrere a strumenti di autoritarismo obsoleto per stimolare un percorso di crescita. Dal prossimo 1° settembre avremo meno sostegno scolastico in tutte le scuole, meno classi nei piccoli Comuni le scuole si troveranno nell'impossibilità di pagare le supplenze. Quali Regioni - e penso al problema del Sud evocato dal Presidente del Consiglio più volte in questi giorni - e quali famiglie più povere saranno in grado davvero di rispettare quanto indicato nella Costituzione, ovvero che i capaci e i meritevoli avranno nella scuola gli strumenti opportuni per emergere? emergere? Se si vuole parlare di università e di cultura, mi basta leggere quanto la vostra maggioranza ha approvato nelle osservazioni. Secondo la maggioranza della Commissione pubblica "In relazione all'università si invita la Commissione bilancio a segnalare, nella relazione che si accinge a presentare in Assemblea, il carattere inderogabile del fabbisogno indicato, anche al fine di recuperare il taglio di 700 milioni di euro sul fondo di finanziamento ordinario previsto a partire dal 2010". Ovvero, come ha detto il presidente della CRUI, nel 2010 le università migliori, anche in questo caso si parla di merito, saranno al fallimento

pur riconoscendo il verificarsi in passato di episodi di cattiva gestione, si deplora il mancato reintegro del FUS nel 2009, tanto che per coprire la vergogna,

tanto più che l'investimento culturale deve essere considerato una scelta di fondo e non una scelta improduttiva. Infine, la ricerca continua ad essere il fanalino di coda in Europa per l'Italia senza alcuna incentivazione.

la strategia dei Governi di altri Paesi - cito per opposti riferimenti politici la Francia e la Spagna - è stata ad esempio quella di investire in maniera fattiva nei saperi, nei saperi, nella consapevolezza che la competitività dei nostri giovani si misurerà sulle loro conoscenze, sulle loro abilità e sulle loro professionalità. Questa è la strada che hanno percorso altri Governi (quella che ha intrapreso il nostro Governo è esattamente l'opposta, ovvero di fare dell'università, della ricerca, della scuola e della cultura il luogo del saccheggio alle risorse), è la strada che il nostro Governo, stoltamente e incomprensibilmente, ha deciso di non percorrere. Signor Presidente, l'anno scorso il DPEF era il documento di avvio programmatico dell'attività di politica economica del Governo e abbiamo tutti salutato, per lo meno dalla mia parte politica, un DPEF per la prima volta leggero, che non era un grosso libro dei sogni e soprattutto che avviava ad una manovra triennale che ci ha consentito, il 15 settembre, con il fallimento della Lehman Brothers, di non trovarci con i conti aperti. Il Documento di programmazione economico-finanziaria è storicamente e strutturalmente complesso, perché incrocia dati di economia reale e di finanza pubblica e li allinea

che costituisce un'importante spinta innovativa rispetto ad una cultura amministrativa rimasta immobile per 150 anni, dall'Unità d'Italia - lo abbiamo ricordato quando in quest'Aula abbiamo approvato la nuova legge sulla finanza pubblica - il Documento di programmazione economico-finanziaria sarà sostituito con la Decisione quadro di finanza pubblica. La riforma è nata dalla necessità di adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica ad esigenze determinate dai recenti cambiamenti istituzionali e dalle condizioni dei conti pubblici. Indubbiamente il Documento di programmazione economico-finanziaria che oggi esaminiamo riflette la grave crisi economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti con il fallimento della Lehman Brothers ed estesasi a tutta l'economia internazionale. La caduta degli scambi internazionali e la riduzione degli investimenti hanno avuto, com'è noto, un forte impatto sull'attività produttiva, stante stante la propensione all'esportazione delle imprese nazionali e il notevole peso dell'industria manifatturiera sul valore aggiunto. Lo scenario internazionale è mutato irreversibilmente e ovviamente l'impatto

Rimane dunque un'elevata incertezza sulle prospettive economiche, anche se iniziano a manifestarsi i sintomi di una timida ripresa. Va dato atto, allora, al Governo di avere agito fino ad oggi con cautela e lungimiranza, garantendo innanzitutto quella stabilità finanziaria che ha consentito al sistema bancario di superare l'impatto negativo della crisi internazionale. Le linee generali del DPEF mettono al centro della politica economica gli investimenti in capitale umano e infrastrutture. La strategia adottata può essere definita in due tempi: un primo intervento per fronteggiare la crisi e tamponarne gli effetti e un secondo per sviluppare l'economia e risanare la finanza pubblica. Il DPEF individua tre obiettivi: la stabilità di bilancio pubblico, la coesione sociale e il credito alle imprese. Nel primo capitolo del Documento il Governo conferma l'impegno di portare i conti verso il pareggio di bilancio e l'obiettivo di una costante riduzione del rapporto debito-PIL non appena la ripresa sarà consolidata. E, come affermato nel DPEF, «il Governo intende agire per trasformare l'attuale crisi in un'opportunità di sviluppo e di rilancio per l'economia italiana, e più in generale di progresso sociale per il Paese». Il Documento ipotizza una ripresa a partire dal 2010. Tali previsioni sono state confermate anche dal rapporto ISAE presentato lo scorso 23 luglio, che evidenzia una ripresa già a partire dal terzo trimestre di quest'anno. inoltre, viene evidenziato che il Governo ha stanziato contro la crisi, senza considerare gli interventi a favore del settore bancario, risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011. A questo si aggiungono 16 miliardi di finanziamenti alle infrastrutture. Le misure anticrisi adottate partire dal 2008 hanno puntato ad aumentare la fiducia tra gli operatori e ridurre l'incertezza, nonché ad aumentare l'efficienza del sistema. Al fine di realizzare il quadro programmatico, il Documento precisa che si interverrà con una azione di contenimento della spesa primaria corrente e con misure che non comportino un incremento della pressione fiscale

*(PD)*. Signor Presidente, stasera discutendo di mozioni abbiamo parlato anche degli impegni internazionali; abbiamo sottolineato l'importanza che il nostro Paese segnali in maniera efficace, significativa e credibile la propria presenza nello scacchiere internazionale.

Faccio questa premessa perché nel DPEF in discussione esiste un'espressione che è un capolavoro di sintesi; peccato che sia terribilmente laconica. A proposito della difesa si dice: «di avere preso misure concrete». Questa espressione non vuole dire niente, non solo perché la concretezza va misurata sulla base di un'elencazione e di una sottolineatura puntuale e specifica, ma anche perché poi nel corpo dello stesso DPEF non si trova niente.

- a mio giudizio questo significa ce l'ha - le chiederei di cercare di contestualizzare in maniera più coerente e, quindi, meno schizofrenica l'attenzione di tipo finanziario e di tipo legislativo da riconoscere al settore della difesa nel momento in cui il nostro Paese è impegnato in ben 32 missioni internazionali. A fronte di questo lievitare delle esigenze e di questo ingigantimento dei bisogni ci sono stati e ci saranno invece tagli lineari che incidono direttamente non solo sul reclutamento e sulla manutenzione, ma addirittura anche sull'addestramento. Non si può andare avanti così. Non si può, come sta accadendo proprio in questi giorni all'interno del Governo, pontificare assumere l'atteggiamento dei difensori dei cosiddetti così - retoricamente i nostri militari vengono definiti ragazzi - dichiarando di volersi preoccupare delle loro condizioni di vita e della loro stessa incolumità, quando poi nella concretezza dei fatti non si fa assolutamente niente; quando poi si tolgono i quattrini; quando poi si demolisce un modello di difesa tagliando, senza alcun tipo di giustificazione, ben 41.000 unità; quando, come accennavo prima, ma soprattutto come molto più autorevolmente di me hanno detto Capi di Stato maggiore di Arma, ne risentono la stessa preparazione e lo stesso addestramento. Allora, se questi cinque minuti di intervento, signor Presidente, possono avere un senso, io li indirizzo, con tutto il rispetto per gli altri presenti, al rappresentante del Governo. A lui chiedo che nel DPEF, oltre a queste quattro paroline che non dicono niente, possa essere inserita una effettiva azione di implementazione a beneficio della Difesa e prevista una posta prevista una posta di bilancio grazie alla quale poter potenziare la cosiddetta difesa passiva, che è ancora carente e che di di fatto non è stata in grado di impedire che anche l'altro giorno un nostro militare morisse sul campo. Visto che noi vogliamo, come Paese civile ed occidentale, svolgere la nostra politica estera, facciamola

Governo, la discussione in corso oggi in quest'Aula sul Documento di programmazione economico-finanziaria è per molti versi l'ennesima occasione mancata. Ancora una volta, a fronte della peggiore crisi economica e finanziaria che abbia colpito il nostro Paese e l'insieme delle economie dei grandi Paesi industrializzati, il Governo si limita a registrare l'esistente, senza indicare alcuna strategia capace di invertire lo stato delle cose. Deve passare la nottata. Questa sembra ormai essere l'unica vera opzione programmatica perseguita dal Governo Berlusconi e, soprattutto, dal ministro Tremonti. Ma mentre passa la nottata, la crisi ogni giorno si fa più grave: un recente rapporto sul mercato del lavoro elaborato dal CNEL evidenzia un quadro estremamente drammatico della capacità di tenuta occupazionale nel nostro Paese. Secondo il CNEL, ma non solo, nel 2009 assisteremo alla scomparsa di mezzo milione di posti di lavoro, che andranno a sommarsi alle varie centinaia di migliaia già persi nel 2008, portando il dato tendenziale di disoccupazione - per il 2009 - tra l'8 ed il 9

In questo scenario, che registra una perdita cumulata del PIL al primo trimestre del 2009 pari a meno 5,9 per cento in termini reali, già largamente superiore alle contrazioni registrate nelle due più gravi recessioni che abbiamo subito dal dopoguerra

l'Esecutivo ancora una volta evita una discussione di merito sulla crisi, come più volte richiesto da noi, capace di delineare alcune opzioni programmatiche utili alla fuoriuscita dalla stessa. Ma non solo: ancora una volta, si costringono le Aule parlamentari a discutere in ritardo, frettolosamente ed in maniera disomogenea. Con la riapertura a settembre delle imprese molte delle questioni verranno al pettine, non ci si potrà nascondere dietro gli annunci o le false promesse: penso alle mancate misure a favore del credito, laddove i provvedimenti del Governo per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese si sono rivelati nei fatti assolutamente inadeguati, e penso al fatto che non si è voluto affrontare il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione dalle attuali 52 a 104 settimane, come più volte richiesto dall'opposizione e da grande parte del movimento sindacale. Un mancato prolungamento che potrà avere drammatiche conseguenze sulla tenuta del nostro sistema industriale e determinare un vero dramma sociale per tanti lavoratori e lavoratrici. Non si è voluto intervenire a favore dei tanti giovani precari, che hanno subito per primi la crisi, con uno strumento universale e straordinario di sostegno al reddito, come più volte il Partito Democratico ha richiesto, ma addirittura si è tenacemente lavorato per il blocco dei processi di stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, quei processi di stabilizzazione previsti e avviati dalle finanziarie del Governo Prodi. Fortunatamente, in merito ai precari della pubblica amministrazione e della scuola, grazie ad una dura battaglia parlamentare e sindacale siamo riusciti ad espungere le parti più gravi dei provvedimenti promossi dal ministro Brunetta, ma siamo ancora molto preoccupati in quanto le misure previste dalla legge n. 133 del 2008 - in ordine alle norme per il *turnover* ed ai vincoli di bilancio - rischiano di rendere estremamente complessi i processi di stabilizzazione. Inoltre, un pronunciamento ufficiale. In sostanza, ci troviamo di fronte all'ennesima occasione mancata, sia per il DPEF quanto in merito al cosiddetto decreto anticrisi, strumento quest'ultimo che forse neanche potremo discutere ed emendare e che sicuramente per chiamarlo "anticrisi" bisogna mettere mano a grandi dosi di fantasia e, mi sia concesso, di sfacciataggine. Un'occasione mancata per un serio dibattito parlamentare, ma ancora di più l'ennesima occasione mancata per il Paese e per le lavoratrici e i lavoratori italiani.

e la percentuale di spesa pubblica per la formazione in rapporto alla spesa pubblica totale per i servizi, dato che già fornisce, peraltro, una indicazione su come eventualmente ottenere delle risorse aggiuntive per università, scuola e ricerca attraverso un riorientamento della spesa pubblica.

Vengono indicate alcune misure che il Governo sta già affrontando, che ha già in cantiere e che saranno approvate nei prossimi mesi. Infine, il DPEF contiene l'indicazione molto corretta, puntuale e onesta delle risorse necessarie. Credo che l'onestà

Riassumo l'ordine degli interventi attorno a questi tre principi chiave: merito, responsabilità, uso intelligente delle risorse pubbliche. è, tra l'altro, un passaggio molto importante che mette in crisi alcune polemiche demagogiche scatenate dall'opposizione, e cioè l'impegno a proseguire le assunzioni dei precari della scuola. Voglio qui ricordare quanto invece l'opposizione ha sostenuto in Commissione, ovvero la necessità di tagliare di un anno il percorso del nostro sistema scolastico. Dico soltanto che una misura di questo tipo, che evidentemente riprende quanto già Berlinguer aveva a suo tempo tentato di realizzare, significherebbe la cancellazione di 80.000 posti di lavoro, e dunque la drammatica scomparsa dalla scena di tutto il precariato italiano. Concludendo, credo che ci siano alcuni passaggi che debbono essere sottolineati con forza. L'università, in particolare, ha bisogno di un investimento nell'eccellenza, in quelle

in quei progetti di ricerca strategici per lo sviluppo del nostro Paese. La scuola ha bisogno di una riforma coraggiosa e radicale del reclutamento, ha bisogno di una differenziazione meritocratica dei salari, ha bisogno di una valutazione dei risultati dei singoli istituti. La prossima finanziaria dovrà essere conseguente. è tracciata una *road map* molto interessante. Per l'università occorre trovare le risorse che nel Documento vengono puntualmente indicate. Devono essere realizzate, a partire dal prossimo autunno, le grandi riforme del reclutamento e della *governance*. che compito del Parlamento, e della maggioranza in particolare, debba essere quello di aiutare il Governo a trovare le risorse necessarie per far realmente decollare il nostro sistema di istruzione e di e di ricerca in modo che sia finalmente competitivo con quello dei principali Paesi europei. Qualche indicazione importante emerge *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, nei pochi minuti a disposizione intendo affrontare un aspetto rilevante ed importante: le politiche per il Mezzogiorno. Nel DPEF è completamente assente ma questa non è purtroppo una novità da parte dell'attuale Governo - qualunque misura di sviluppo in favore del Mezzogiorno, area già fortemente penalizzata dai provvedimenti adottati dal Governo nel primo anno di legislatura. Nel corso del mio intervento citerò il sostanziale svuotamento del FAS, il taglio delle risorse destinate alle infrastrutture e il blocco del credito d'imposta per gli investimenti nelle Regioni meridionali. In questi giorni, dopo silenzi e disattenzioni, è scoppiata - si può proprio dire così - la questione meridionale. Mi verrebbe da esclamare: era ora! Ma qualche timore che le ferie di agosto mettano la sordina c'è; qualche preoccupazione che si tratti solo di effetti speciali o di propaganda per zittire o tranquillizzare qualche alleato turbolento c'è. Non è sfiducia preventiva nei confronti del Governo e della maggioranza: è mera osservazione dei fatti, degli scellerati atti che fin qui sono stati compiuti. È da più di un anno che Berlusconi e il suo Governo hanno ignorato il Sud, così come hanno ignorato le denunce e le proposte giunte dal Partito Democratico e dall'opposizione. Ricordo solo, ad esempio, la mozione sulle infrastrutture nel Mezzogiorno, bocciata in quest'Aula qualche mese fa. Non solo, tutta l'azione dell'Esecutivo, puntualmente sostenuto dai parlamentari della maggioranza, settentrionali e meridionali, è stata finalizzata a penalizzare le speranze di sviluppo del Mezzogiorno e a privilegiare,

la quota nazionale (26-27 miliardi) è andata in fumo, usata come un bancomat per tamponare emergenze, per tappare buchi in bilancio, per rispondere alle più svariate esigenze, molte delle quali provenienti dal Nord del Paese. Abbiamo denunciato e avanzato proposte da questi banchi, senza farci mai suggestionare da ipotesi di partiti del Sud da contrapporre a partiti del Nord. Siamo fermamente convinti che quella meridionale, così come ci hanno insegnato Giustino Fortunato e Manlio Rossi Doria, sia una grande questione nazionale e che in questo modo vada affrontata. Si tratta di un grande confronto che necessariamente dobbiamo aprire fra di noi, in Parlamento: è la politica che si deve riappropriare della questione meridionale. La politica deve essere in grado di dare un pensiero, filoni culturali, strategie e proposte. Su questo terreno mi pare che le parole scritte su «Il Mattino» di Napoli dal senatore Quagliariello possano rappresentare un terreno di confronto, che almeno compensa certi sconfortanti atteggiamenti espressi da alcuni Ministri del Nord che tendono ad assimilare il giudizio al pregiudizio e definiscono il Sud «piagnone e sprecone». Ricominciamo dal confronto, ma per favore non mettete sul campo minestre ormai inacidite, riscaldate e trucchi da prestigiatori: non vi venga in mente di riproporre la Cassa per il Mezzogiorno o il Ministero per il Mezzogiorno. Questo leggiamo nelle dichiarazioni. La prima ipotesi è uno strabico ritorno al passato, a cinquant'anni fa, e quindi non è una grande idea, e il Ministero ci sembra soltanto un modo per sistemare qualche scontento in vista del rimpasto, mini o maxi, prossimo venturo. E non venite a raccontare al Paese e al Parlamento che sbloccherete i fondi FAS. Quali? Quelli già assegnati? Quelli dati all'Abruzzo? O si ripristinano da altre fonti di finanziamento quei fondi o sarete costretti a fare un altro scippo, cioè a prendere i fondi del FAS delle Regioni e accentrarne la gestione. Se si vuole riparlare seriamente del Sud si riparta da una seria analisi delle condizioni che vive oggi quell'area. Vado di fretta, quindi ricordo soltanto che esiste il rapporto dello SVIMEZ che dice tante cose sul Sud. Tale rapporto dice che il Sud si sta svuotando e soprattutto si sta svuotando di giovani: un laureato su due del Sud va altrove. Bisogna ricominciare con serietà e concretezza. Abbiamo presentato alcune proposte

la piena operatività degli strumenti di automazione e di incentivazione, quale il credito d'imposta sugli investimenti per il Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e degli appesantimenti amministrativi concessi al meccanismo della prenotazione. Ecco, da queste cose serie e concrete si deve ricominciare.

sulla base dei dati che ci offre il Documento di programmazione economico-finanziaria, affinché le politiche pubbliche, che moltiplicano i centri di intermediazione della pubblica amministrazione senza creare nuovo benessere per i cittadini, siano messe a valutazione.

quindi convinti che il settore pubblico abbia bisogno di una chiara e verificabile presenza di indicatori di *performance,* in modo da

In questa direzione si sono mosse le riforme onestamente avviate in questo primo anno di legislatura, se vogliamo parlare di questa legislatura. La vicenda del federalismo fiscale è sicuramente una riforma e le riforme non si attuano in un giorno: è un processo in atto che punta a produrre effetti di responsabilizzazione dei centri di spesa. Il riordino del nostro *welfare* verso un nuovo modello di Stato sociale e la riforma della pubblica amministrazione: tutti fattori di inefficienza, per ammissione di tutti, che hanno pesato nella formazione dell'attuale distanza tra i tassi di crescita del nostro Paese al netto della crisi del momento e quelli degli altri Paesi più avanzati. Vi è poi il capitolo del Sud e il connesso tema e il connesso tema dell'utilizzo dei fondi FAS, che tengono banco in questi giorni e hanno tenuto banco in questi mesi. Sul Sud non possiamo dividerci - lo dico anche ai colleghi dell'opposizione e agli amici della Lega - tra coloro che ragionano sul presupposto che al Sud i soldi ci sono, ma si spendono male e quanti, in ragione di tale assunto, archiviano la complessa questione derubricandola al massimo ad una disputa che nasconde pure lotte di potere. Bisogna ammettere che c'è un'area del Paese - non lo scopriamo oggi - che, peraltro nell'ultimo decennio, quindi sfiorando trasversalmente tutti i Governi, non ha recuperato il suo svantaggio strutturale e produttivo. Questo è il dato di fatto, e gli indicatori indipendenti ce lo confermano. questo è il punto di osservazione che chiama in causa anche le responsabilità dei governi regionali - due Quadri comunitari di sostegno (1994-1999 2001-2006) che avrebbero dovuto raggiungere obiettivi di coesione tra le Regioni dell'obiettivo 1 e le altre Regioni più avanzate d'Italia e d'Europa. Bisogna sottolineare che l'intervento europeo ha fallito spesso per la disarticolazione dei piani operativi redatti e gestiti dalle Regioni, ma va pure notato con onestà intellettuale che quello europeo alla fine è stato un intervento non aggiuntivo, bensì sostitutivo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno d'Italia. è una questione di qualità della spesa, di coordinamento della stessa. Sarebbe il caso, signor Vice Ministro, di non indulgere oltre perché, mentre parliamo, le Regioni dell'obiettivo 1 si apprestano ad attuare i programmi per il 2007-2013 che stanno per mobilitare una massa imponente Chiediamo al Governo di dare corso a quella intesa con le Regioni del Mezzogiorno che metta insieme tutte le risorse disponibili per obiettivi di potenziamento del sistema produttivo e infrastrutturale. C'è però ugualmente - lo dobbiamo ammettere - una questione quantitativa. È giunto il momento che si faccia chiarezza sull'effettivo impiego delle risorse FAS e sul rispetto del vincolo che vuole che l'85 per cento dello stesso fondo sia destinato alle aree del Mezzogiorno. che il Paese vive una sua illusione se pensa di risolvere la questione dell'accrescimento della competitività senza il Mezzogiorno, come pure sarebbe una tragica illusione pensare di affrontare i problemi meridionali senza un solido ancoraggio alla politica nazionale.

di intervenire. Il motivo è legato ad una manifestazione programmata per domani, alle ore 12, nella Sala Nassirya. Si tratta di una conferenza stampa aperta a tutti i senatori, in particolare a coloro che hanno firmato un'interrogazione ed una lettera al Presidente del Consiglio sul caso dell'italiano - il trentino Enrico (detto Chicco) Forti - detenuto nelle carceri di Miami, negli Stati Uniti, ormai da 10 anni con l'accusa di aver ucciso un uomo (che lui dice di non aver ucciso), a cui è seguita una pesante condanna all'ergastolo. Forti ormai da 10 anni chiede semplicemente non la grazia, non di tornare in Italia, ma di poter riaprire il processo, in quanto ha in mano prove determinanti (le aveva anche all'inizio, ma non gliele hanno lasciate presentare) per dimostrare la sua estraneità al

documentare questa sua legittima aspirazione: l'istanza, rivolta alla Corte federale, di poter riaprire il processo. Proprio oggi è giunta anche una toccante testimonianza, un suo messaggio audio dal carcere duro di Miami, con il quale fa pervenire a tutti noi, in viva voce, la sua richiesta di essere ascoltato e nuovamente L'invito è rivolto a tutti, non solo alle persone di buona volontà presenti nell'emiciclo in questo momento, ma anche ai colleghi che tenacemente sono negli uffici a lavorare. In ogni caso, domani mattina faremo un passa parola perché a volte la solidarietà ha un peso maggiore se maggiore è la partecipazione della gente.

la scuola "Giovanni Falcone", un plesso scolastico che insiste nel quartiere San Filippo Neri di Palermo (più noto come quartiere ZEN).

chiedo alla Presidenza del Senato di sensibilizzare il Ministro dell'interno per fare in modo che quella scuola venga considerata come obiettivo sensibile.